la Commissione industria, commercio, turismo ha esaminato in cinque sedute e per diverse ore l'Atto Senato n. 1427. Dopo la relazione e il dibattito in discussione generale, con le relative repliche, una volta iniziata l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, non si è potuto procedere oltre quelli riguardanti l'articolo 5. A fronte dell'illustrazione di circa 30 emendamenti, su un totale di 230 presentati, la Commissione ha ritenuto necessario interrompere l'esame, a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione per il seguito dell'esame. In questa maniera, la Commissione non ha potuto procedere ad un completo ed esaustivo esame di un provvedimento complesso e articolato, non essendo in grado, in ultima analisi, di assolvere per completo alla sua funzione referente. Si ritiene infatti che l'esame di un testo di tale portata e complessità avrebbe necessitato della disponibilità di ben più ore di lavoro. Per tali ragioni, signor Presidente, la Commissione ha ritenuto opportuno rimettere il testo all'esame dell'Assemblea. In relazione a quanto riferito dal senatore Maninetti, il disegno di legge n. 1427, non essendosi concluso l'esame della Commissione,

Io sono pregiudizialmente contrario alla discussione perché le disposizioni, signor Presidente e illustri colleghi, principalmente proprio quella dell'articolo 1 del decreto-legge, a nostro avviso sono farraginose, demagogiche e fuorvianti. Sono fuorvianti in specie di una presumibile ed auspicabile evoluzione in senso liberale del mercato. Signor Presidente, com'è noto, questo decreto ha finito per essere presentato e titolato all'opinione pubblica come un intervento del Governo a favore del consumatore, per garantire un mercato trasparente e, significativamente, nella titolazione più abusata ed usata, per far costare meno il servizio di telefonia mobile. mobile. È tuttavia successo che durante l'*iter* parlamentare, e puntualmente nelle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, è stato osservato che il minor costo delle tariffe telefoniche, così come presumibilmente

minor tassazione ad imposizione diretta nei confronti degli operatori di telefonia. A questo punto, osservato questo nelle Commissioni, il Governo dichiara...

Il telefono deve costare meno, se costa meno ci sarà un minor fatturato, se c'è un minor fatturato ci sarà un minor gettito IVA. E allora la Commissione bilancio domanda al Governo: di cosa si tratta? Dobbiamo prevedere nel bilancio la minor rinvenienza del gettito fiscale. A questo punto, il Governo, Presidente e colleghi, dichiara (leggo testualmente): «si rileva che il venir meno del contributo di ricarica nei servizi di telefonia mobile a credito prepagato non comporta non comporta sostanziali effetti in termini di gettito». E segue: «determinando» (la diminuzione del costo) «il concomitante effetto da un lato della ristrutturazione delle tariffe». Lo dichiara il Governo: non cambierà nulla, perché le tariffe terranno conto della diminuzione del costo e quindi recupereranno il minor pagato. Allora, se è lo stesso Governo a dire che le tariffe aumenteranno, a cosa serve il decreto? Serve, a nostro avviso, a spacciare un intervento inutile e dannoso per un regalo ai cittadini. *(Brusìo)*.

C'è di più: il provvedimento - il linguaggio parlamentare a questo punto ci consiglierebbe di dire almeno ultroneo - è a mio avviso avviso inutile, perché nel nostro ordinamento esiste già un decreto legislativo, il n. 259 del 2003 (voglia il Governo prendere nota perché probabilmente non l'ha letto), che è il codice delle comunicazioni elettroniche, che all'articolo 71 demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare che siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori informazioni trasparenti,

nella quale si esprimevano preoccupazioni sull'argomento. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, congiuntamente a quella per le garanzie nelle telecomunicazioni, il 16 novembre aveva esitato un documento d'indagine che condannava la situazione. Ci domandiamo: perché, se c'era un documento di condanna, non sono state già allora comminate le sanzioni? Perché la necessità di un provvedimento legislativo? Il quesito è: siete liberali o siete statalisti?

non lasciando la libertà agli operatori e quindi facendo venir meno dei gradi di libertà del mercato. Ma c'è anche - ed è la questione atipica sospensiva - un'altra libertà che con questo provvedimento si va a ridurre. Presidente, una libertà ben più importante, perché il Governo, in modo ripetuto, abusato e violento, sta riducendo la libertà del Parlamento.

epocale, strabiliante, in soli cinque giorni? Noi stiamo discutendo un provvedimento importante, strabiliante ed epocale in cinque giorni. Si parla sempre di rispetto della Costituzione e invece, introducendo di fatto un monocameralismo, la stiamo violando; alla faccia dell'invocata perfezione del sistema! Vogliamo ricordare che al momento della tornata referendaria, nella quale si discuteva di asimmetria parlamentare, da quella parte politica sono state, nelle piazze e in televisione, invocate le giuste ragioni dei Padri costituenti, sostenendo che il bicameralismo perfetto in Italia era una garanzia di democrazia. In questo momento, invece,

è uno strumento procedurale dedotto dal Regolamento ma non regolamentato. Non solo, ma nel momento in cui se ne discusse, si pensava che potessero e dovessero esserne conforto alcuni elementi, quali l'urgenza, la sufficiente trattazione e un eccesso di emendamenti per cui doveva essere salvaguardato, al di là della posizione della questione di fiducia, il diritto del cittadino a decidere

È contro il Paese non discutere sui miliardi di euro che ipoteticamente derivano dalla definitiva introduzione della disposizione in esame. La La mia proposta è quella di procedere invece attraverso una formulazione atipica della questione sospensiva, e cioè nella trasformazione del decreto in disegno di legge, nella stessa veste con la quale ci proviene dalla Camera dei deputati, esaminarlo con procedura di estrema urgenza e consentire quella discussione sulle leggi che ormai, Presidente, secondo me e secondo noi da troppo tempo manca da quest'Aula. Noi in quest'Aula non discutiamo più di leggi. Ho paura, Presidente, che

è un decreto-legge che va al di là del titolo, ancorché ricco, perché se lo leggiamo si parla di tutela per i consumatori, di promozione della concorrenza, di sviluppo delle attività economiche, di nascita di nuove imprese, ma in realtà esso contiene norme che nulla hanno a che vedere con con il titolo, e che possiamo vedere riassunte invece nell'intitolazione dell'articolo 13, introdotto con il maxiemendamento del Governo, laddove l'Esecutivo ha dovuto svelare l'unico testo che il decreto-legge contiene: norme sulla pubblica istruzione, istruzione, sulla rottamazione, sulla pubblicità immobiliare, sulle concessioni TAV, sul nostro ordinamento fondamentale in materia di procedimenti amministrativi. Vi sono poi aspetti, colleghi, che riguardano chiare ipotesi di invadenza e di invasione della competenza statale nelle competenze regionali, e mi meraviglio

contiene norme che invadono la competenza regionale e che vengono coperte dal cappello della tutela della concorrenza, competenza statale, la quale dovrebbe quale dovrebbe far superare ogni dubbio sul modello di competenze che - ricordo - non è stato disegnato dal centro-destra centro-destra ma dal centro-sinistra e che noi ci siamo sforzati per cinque anni di Governo, e non senza sofferenze, di rispettare. Con la scusa della tutela della concorrenza si dettano, invece, norme che invadono la competenza regionale. Ma vi sono

per le norme regionali ma sono chiaramente di competenza concorrente tra Stato e Regioni in base al terzo comma dell'articolo 117 della le norme in materia di istruzione professionale, quali quelle reintrodotte espressamente nel decreto‑legge attraverso il recupero degli istituti professionali. Sono ‑ ve lo ricordo ‑ competenze esclusive ancorché in un quadro più generale dettato dallo Stato. Ieri, Presidente, si è discusso delle questioni relative ai presupposti quindi non le ripeto, ma anche queste sono questioni di carattere costituzionale. Molte norme del decreto‑legge in esame non sono entrate in vigore. Vi sono norme manifesto come l'articolo 9, battezzato "la norma delle imprese in un giorno". È chiaro, però, che si tratta di perché, se non modifichiamo quanto c'è prima della concessione dell'autorizzazione, è evidente che le imprese in un giorno rappresentano un sogno, un manifesto, un'utopia e certamente non una realtà che possa formare oggetto di un decreto-legge.

segnale molto grave della mentalità centralista e statalista del Governo. Voglio soffermarmi brevemente su un altro in particolare ai colleghi che hanno qualche cognizione giuridica e naturalmente a quelli che considero giuristi (magistrati, avvocati, docenti universitari, chi abbia esperienza giuridica),

blindato, con un maxiemendamento, una norma che scardina un principio fondamentale di questa legge; principio, direi, ancor più fondamentale

sotto il Governo Berlusconi), poiché si è ritenuto che questa fosse una norma di civiltà; la norma di civiltà prevedeva che la pubblica amministrazione potesse provvedere alla revoca di provvedimenti amministrativi solo in presenza della sopravvenienza di interessi pubblici, ovvero nel caso in cui vi fosse ragione di valutare diversamente la presenza di interessi pubblici. Naturalmente, questa revoca avrebbe questa revoca avrebbe determinato le conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento in via generale, cioè risarcimento dei danni a carico della pubblica amministrazione, costituiti sia dal cosiddetto danno emergente, cioè dai costi che il soggetto privato aveva sopportato una volta ottenuto il provvedimento di concessione o autorizzazione, sia il cosiddetto lucro cessante, cioè la prospettiva di guadagno che con la revoca veniva meno. Ebbene, poiché il decreto-legge prevede la revoca delle concessioni TAV, allora il buon ministro Bersani, o meglio, per lui sicuramente il ministro Pecoraro Scanio o il ministro Di Pietro (e mi meraviglio che il ministro Di Pietro, così sensibile alle ragioni del diritto, poi strappi le regole giuridiche quando questo gli conviene per ragioni politiche o per ragioni del suo Ministero) prevedendo che la

che i danni sono commisurati solo al danno emergente, poi costruendo una formulazione barocca per cercare di tirare dentro anche il privato e dire che, se il privato era in grado di conoscere che l'interesse pubblico era prevalente, allora avrà un danno ridotto o addirittura nessun danno. Ma vi è di peggio: proprio perché questa norma è funzionale alla normativa sulla revoca TAV, il legislatore, o meglio il Governo, ha ritenuto di stabilire la retroattività di questa normativa, venendo a far cadere uno dei princìpi cardine del nostro ordinamento giuridico. Alla faccia del rispetto delle regole, alla faccia della

a quest'arroganza del potere da parte del centro-sinistra, del Governo e di una maggioranza che nemmeno alza un alito di critica verso queste norme che gridano vendetta. per favore.

La questione giuridica è da inquadrare nella revoca delle concessioni che all'inizio degli anni '90 l'ente Ferrovie dello Stato fece alla società TAV (Treno ad alta velocità) per la progettazione e la costruzione di oltre 1.000 chilometri di nuove linee ferroviarie ad alta velocità. La TAV mobilitò, per tali adempimenti, contraenti generali come l'IRI, l'ENI, la FIAT e la Montedison e altre grandi imprese, tutte quotate in borsa. Gli azionisti delle imprese contraenti della TAV Spa, che hanno ricevuto la revoca da questo decreto, hanno ricomprato le azioni dall'IRI facendo ricorso al mercato finanziario regolamentato. La revoca delle concessioni, pertanto, colpisce l'affidabilità dello Stato su due fronti: quello verso l'autonomia negoziale con cui i contraenti generali hanno stipulato le convenzioni accessive alle concessioni; quello verso gli azionisti, piccoli risparmiatori, che hanno comprato azioni dell'ex IRI poste sul mercato a seguito del processo di privatizzazione che ne è derivato negli anni '90, quando era primo ministro Prodi. La violazione dell'articolo 41 della Costituzione è rilevabile sotto diversi profili. Il primo: le concessionarie, come detto, sono imprese che hanno stipulato in autonomia negoziale convenzioni accessive alle concessioni. Tutte hanno assunto obbligazioni, elaborato programmi industriali sulla scorta delle stesse convenzioni. La revoca e la conseguente estinzione del rapporto concessorio costituisce una lesione del tutto irragionevole di iniziative poste in atto in forza di legge e ad iniziativa del concedente. I vincoli e le limitazioni che sono state prodotti non erano valutabili *ex ante* perché inesistenti e perciò del tutto imprevedibili. È palese, quindi, la violazione del principio dell'affidamento. La Corte costituzionale ha più volte fatto riferimento a tale principio, ad esempio nella sentenza del 19 marzo-4 aprile 1990, n. 155, dove si legge connesso alla libertà di iniziativa economica privata, da garantire, come è ormai *jus receptum*, non solo nel momento iniziale, ma anche durante il suo dinamico sviluppo, al quale appunto, si ricollega il ricordato principio». Qui, con questo decreto, non solo si è inciso su situazioni poste in essere dalla legge, ma anche su contratti, ossia le convenzioni stipulate con la TAV in base a concessioni dell'ente Ferrovie dello Stato, allora amministrazione statale. Costituzione riguarda le società che hanno acquisito il capitale a seguito di dismissioni da parte di enti pubblici statali come l'IRI. Qui la violazione dell'affidamento e del principio di certezza del diritto, e con esso dell'articolo 41 della Costituzione, è ancora più evidente in quanto si contravviene ad un affidamento ingenerato in base ad un'iniziativa legislativa da cui sono discesi poi rapporti contrattuali tra privati di diversa specie. E veniamo ora al terzo profilo: è violato il contenuto essenziale dell'iniziativa economica privata, perché l'intervento sulla legge è di tale entità da cancellare il contenuto essenziale del diritto alla iniziativa economica in essere ed è da segnalare, inoltre, che tale principio dell'affidamento è violato anche nella materia assicurativa, disciplinata dall'articolo 5, per la parte in cui si modificano le polizze poliennali con effetto retroattivo, stravolgendo *ope legis* il principio della libera iniziativa economica e della libera organizzazione di impresa. Non va poi sottaciuta la violazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come derivante dalla modifica del 2001 del Titolo V. La materia delle grandi reti di trasporto è materia concorrente, di modo che lo Stato può solo dettare norme di principio e non produrre normativa di estremo dettaglio che di fatto cancella intere tratte ferroviarie già date in concessione, come la Milano-Verona,

Va sottolineata inoltre l'infondatezza della relazione tecnica e quindi della violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che viene dichiarato apoditticamente che nessun onere aggiuntivo è a carico della finanza pubblica. L'idea che gli indennizzi sarebbero compensati dai risparmi attesi dai ribassi d'asta, prendendo a base il costo finale (38 milioni di euro per chilometro) della tratta di Bologna rispetto agli 82 milioni di euro della Firenze-Bologna è molto aleatoria. Rimando infatti ogni considerazione alle affermazioni pubblicate a pagamento dalle imprese interessate su «Il Sole 24 ORE» dell'altro ieri dove vengono denunciate le falsità di tale presupposto in quanto non tengono conto delle rivalutazioni, riserve e slittamenti dei termini registrati, che hanno recuperato ampiamente quel 46,9 per cento di ribasso d'asta acquisito. Non parliamo poi degli oneri per contenziosi che deriverebbero da tale revoca con il rilievo del danno emergente - qui rilevato dallo stesso collega Pastore - che soppianterebbe ampiamente la formula dell'indennizzo dovuto per danno da fatto lecito. Sul piano politico va sottolineata la falsità delle affermazioni che i contraenti generali siano revocati perché inefficienti. A 16 anni dall'affidamento dei tronchi dati in concessione, non è stato ancora dato il previsto finanziamento, ancorché i progetti da realizzare siano pronti. Sicché i lavori non sono stati fatti per la semplice ragione che non sono mai stati dati i relativi finanziamenti. È falso anche che i costi siano fuori mercato, perché la loro congruità è determinata dalla Italferr, società di ingegneria del gruppo Ferrovie dello Stato, assistita da primarie consulenze internazionali. C'è il fondato sospetto di alcune vendette politiche e soprattutto la strana idea di inseguire interlocutori con cui far fare strane cordate di ben note imprese italiane di un certo mondo cooperativo. Al momento rimane la constatazione che: si vìola la norma costituzionale con la lesione del principio di affidabilità, come evidenziato; si cancellano tre tratte primarie dell'Alta velocità nel Nord; nel Nord; si fanno perdere all'Italia - oltre quelli già persi per il ponte sullo Stretto di Messina - più di 2 miliardi di euro di contributi in conto capitale destinati dall'Unione Europea per la realizzazione dei corridoi europei Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam, dei quali le linee revocate sono segmenti. Un capolavoro di imbecillità politica senza eguali in Europa. Complimenti, ma fermatevi qui e fermatevi presto!

provvedimento è stato indubbiamente presentato con cura e abilità alla grande stampa di opinione come il fiore all'occhiello di una volontà liberalizzatrice del Governo Prodi che in realtà secondo la nostra opinione, contiene norme illiberali ed incostituzionali. Il riferimento è chiaramente all'articolo 13, là dove, con un provvedimento di legge, si dispone la revoca di un atto amministrativo consensualmente sottoscritto per realizzare importanti infrastrutture ferroviarie del nostro Paese. Così, se domani - come sembra questo decreto-legge sarà convertito, le tratte dell'Alta velocità Genova-Milano e Milano-Verona-Padova, affidate anni addietro a due *general contractor*, saranno revocate, con notevole pregiudizio per la loro Il Nord evoluto pagherà ancora una volta un prezzo elevatissimo per l'incapacità di un Governo che a parole dice di voler credere sull'infrastrutturazione del Paese e nei fatti si comporta in maniera assai diversa. Le motivazioni politiche sono ben chiare a tutti noi. La maggioranza che sostiene il Governo Prodi non crede al processo di infrastrutturazione del Paese (signor ministro Bersani, magari nella replica ci ricordi qual è l'infrastruttura che, in giacenza dell'attuale Esecutivo, sia stata avviata, accelerata e realizzata nei primi nove mesi di vita del vostro Governo). Non crede all'infrastrutturazione del Paese questa maggioranza, perché è condizionata da Gruppi parlamentari che da anni si battono con tutti i mezzi per impedire che l'Italia sia dotata di infrastrutture viarie e ferroviarie necessarie ad aumentarne la competitività. Quando a Genova venne divulgata la notizia che il Governo aveva revocato la concessione dell'Alta velocità per la tratta Genova-Milano, esponenti qualificati dei Gruppi Verdi e Rifondazione Comunista hanno festeggiato in un noto albergo genovese. Il dibattito di merito, signor Presidente, consentirà di approfondire questi aspetti, così da smascherare talune affermazioni a nostro modo di vedere improprie, false e demagogiche, servite al ministro Bersani a guadagnarsi momenti di popolarità a poco prezzo. Quando egli afferma che le concessioni revocate sulla TAV riguardano infrastrutture non partite, non ancora avviate a realizzazione, sostiene il falso, ben sapendo che, ad esempio, per la tratta Genova-Milano sono già stati spesi 250 milioni di euro. Se il ministro Bersani avesse colloquiato con il suo collega di partito, il senatore Mazzarello, forse avrebbe saputo che lo stesso, nella sua qualità di assessore ai trasporti della Regione Liguria, andò ad inaugurare il foro pilota che costò negli anni addietro più di 120 miliardi di lire.

dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, nonché da tutte le Province interessate al tracciato, e per la quale il bilancio dello Stato ha già speso più di 500 miliardi di vecchie lire. Signor Ministro, mi consenta pertanto di asserire che le sue affermazioni contenute nella pregevole intervista del 30

Quando nel suddetto articolo 13 si legge che il *general* *contractor* può essere risarcito, ma in misura diversa da altri interlocutori (ipotizzando, quindi, una minore protezione di fronte alla legge) chiaramente si vìola l'articolo 3 della Costituzione, che afferma il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Principio, signor Ministro, assolutamente applicabile anche in presenza di leggi provvedimento, cioè di leggi che riguardano qualcosa di specifico, come la problematica in discussione quest'oggi. Ancora, l'articolo 13 vìola la Costituzione laddove ignora che gli articoli 41 e 42 della stessa, tutelando l'iniziativa economica privata, non consentono al legislatore la discrezionalità di intervenire nella contrattazione privata. Siamo in presenza di una legge che interviene a gamba tesa sulle parti che hanno consensualmente stipulato un contratto.

immaginare che due parti private sottoscrivano un contratto che poi può essere messo in discussione da un decreto-legge, tanto più nella situazione - come la nostra - di un Paese evoluto, che fa parte del G8. Decisioni di questo tipo, signor Ministro, sono proprie di Paesi sottosviluppati, nei quali non esiste la certezza dei diritti ed ai quali - come lei sa bene - la SACE, quando interviene a garanzia di un contratto, fa pagare commissioni superiori al 12 per cento, proprio a causa dell'alto rischio esistente

che consente al Governo di intervenire con decreto-legge solo nei casi di urgenza e necessità. Signor Ministro, ma queste due opere di cui oggi revocate le concessioni lei lo sa che sono ferme da quando siete andati al Governo? Le avete messe su un binario morto; non le avete giudicate né prioritarie, né fondamentali, né urgenti. Dopo aver tenuto ferme due opere per dieci mesi oggi volete farci credere che c'è l'urgenza e la necessità di proporne la revoca attraverso un decreto. Mi pare che questo sia un assurdo, com'è un assurdo - e lei dovrebbe saperlo, signor Ministro - che nella convenzione sottoscritta dal *general* *contractor* con la TAV e l'Italferr ci sia un articolo che stabilisce che, in presenza di un disaccordo sul prezzo giudicato da alcuna delle parti non congruo, la TAV, pagando il 3 per cento, può uscire dal contratto prendendosi il progetto. Quindi il Governo, il suo Governo, su sua proposta, anziché scegliere la soluzione maestra e corretta strada amministrativa ha preferito la forza della legge, esponendo l'erario ad un contenzioso che siamo certi supererà il miliardo di euro. Un contenzioso i cui costi futuri, senatore Morando, presidente della Commissione bilancio, non

motivo riteniamo la norma incostituzionale, perché priva di copertura e perché viola l'articolo 81 della Costituzione. E non possono essere di aiuto le considerazioni contenute nella relazione di accompagnamento del decreto, là dove si prevede che revocando la concessione e facendo gare europee si potrà risparmiare il 20 per cento dei conti. Già nel 2000, dei conti. Già nel 2000, signor Presidente, il ministro dei trasporti Bersani ci fece credere una cosa simile. Allora c'era l'ingegnere Cimoli, oggi c'è l'ingegnere Moretti, entrambi grandi professionisti, grandi tecnici, grandi*manager*, dotati di una elevata professionalità, che forniscono, a mio modo di vedere, valutazioni improprie per convincere il Governo a fare quello che sta facendo. Purtroppo allora le Ferrovie bloccarono le opere, furono costrette a pagare sanzioni nell'ordine milioni di euro e non fu realizzata nessuna tratta. Questo accadde nel 2000 e a mio parere accadrà ancora. Il Governo, invece di proporre un provvedimento di revoca, che avrebbe dovuto fare la pubblica amministrazione, stabilisce con norma quanto dovuto anche al privato. Perché tutto questo? Per ignoranza degli estensori della norma? Credo proprio di no, signor Presidente. La mia opinione è che siamo in presenza di una scelta di un Governo che, conscio di non percorre la strada maestra di una revoca, compie una rottura assai grave del sistema. Lo dico riferendomi ai costituzionalisti presenti: siamo in presenza, cari colleghi,

a comitato esecutivo del volere del Governo, come fece già nella finanziaria! È triste, cari colleghi, assistere impotenti ad atti di così elevata arroganza; è triste constatare che nel nostro Paese al cittadino non rimane che confidare su strumenti indiretti come la Corte costituzionale e la Corte di giustizia; è triste, signor Presidente, ed è un sintomo preoccupante del degrado delle istituzioni, constatare

quello che prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente da entrambe le Camere. Questo decreto-legge non solo non contiene misure di straordinaria necessità ed urgenza, non solo presenta un coacervo di norme che nulla hanno a che fare l'una con l'altra, ma è stato anche premeditamente portato all'attenzione del Senato in modo che questo non potesse in alcun modo dare il suo contributo nell'elaborazione di norme - che sono norme legislative - che dovrebbero essere invece affidate alla procedura ordinaria di un disegno di legge. Ricordo che la Costituzione, all'articolo 73, prevede anche che ordinariamente

Non contento di questo, il Governo ha attuato la strategia di allungare i tempi di discussione alla Camera. Mi riferisco al fatto che in Commissione si è arrivati all'approvazione definitiva il 21 febbraio, la bellezza di 21 giorni dopo

alla Camera il provvedimento è stato tenuto nel cassetto. Se quei 16 giorni fossero stati utilizzati per l'approvazione avrebbero consentito due settimane

no, dire al Governo che la facoltà legislativa appartiene alle Camere, che il Senato è disposto ad esaminare un disegno di legge di contenuti analoghi decreto in discussione, in modo tale da poter esercitare le facoltà che la Costituzione e i cittadini gli affidano. Come se non bastasse, questa gravissima violazione di una norma fondamentale dellaCostituzione viene fatta ad un preciso (tacendo quelli più oscuri, nascosti nell'immenso e caotico articolo 13), quello di lanciare un piccolo *spot* di immagine. Dopo le tante brutte figure collezionate dal Governo in tutti i campi, si si è vista l'opportunità di elaborare alcune norme da *spot* commerciale per dare finalmente una buona immagine di sé.

non lo dice per sua semplice congettura, ma traendone la certezza da documenti presentati dal Governo, dalla relazione tecnica del Governo e dalle affermazioni del sottosegretario Lettieri alla Camera, il quale ha detto che la rimodulazione

finzione giuridica. In realtà, i tempi necessari per rendere operativa un'impresa sono esattamente quelli di prima. Anziché fare l'impresa in un giorno, in realtà si vuole fare la legge in giorno e la legge la vuole fare il Governo per conto suo, senza rendere conto né al Senato né al Paese.

Signor Presidente, desidero porre una questione all'attenzione del Senato. La nostra Costituzione, all'articolo 99, prevede il CNEL quale organo di alta consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Il nostro Regolamento, poi, all'articolo 49, commi 1 e 2, disciplina la questione per quanto riguarda il procedimento in Commissione e, all'articolo 98, per quanto riguarda l'Assemblea.

Abbiamo bisogno di migliorare la qualità della legislazione e tutto ciò invece viene meno, soprattutto quando si rafforza il convincimento di un eccesso di potere legislativo imposto dal Governo con un atto fiduciario rispetto al Parlamento. Non siamo nella condizione di emendare nulla. non ci viene permesso nemmeno di presentare ordini del giorno, che non possono essere discussi in Commissione perché il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione industria senza neppure il mandato al relatore Su un provvedimento ritenuto di straordinaria importanza dal Governo, da noi certamente un po' meno rispetto all'impostazione generale, essendo qui in discussione finte liberalizzazioni, mandato al relatore e senza il parere del CNEL, un organo di rilevanza costituzionale. Senza entrare nel merito di disposizioni importanti, signor Presidente, che vanno dalle licenze UMTS alla TAV, dalle questioni assicurative, che riguardano tutti i cittadini, ad altre questioni come quelle dei mutui, noi non abbiamo nulla. Sulla TAV, poi,

non abbiamo visto un atteggiamento di questo genere da parte dell'attuale maggioranza; anzi, allora si richiedeva il parere del CNEL. Ricordiamo bene nella scorsa legislatura gli interventi che venivano posti in questa direzione. direzione. Mi piace sottolineare che non vedo presente il ministro Bersani. Non stiamo facendo liberalizzazioni: stiamo passando dal capitalismo di Stato al capitalismo regionale. Non si affronta il problema vero che è quello delle *multiutility*. Non si affronta il problema delle rendite di posizione.

sta andando in direzione di una cooperazione che gode di vantaggi fiscali e che altera la concorrenza proprio perché usufruisce di vantaggi che devono essere rimossi. signor Presidente, poiché manca un parere tanto autorevole, che in passato veniva sollecitato e che oggi invece viene dimenticato, questo metodo inaccettabile in quanto mortifica il Parlamento su questioni che toccano la vita dei cittadini e chiediamo pertanto che questo parere possa essere espresso.

Presidente, rispondo alle numerosissime argomentazioni messe in campo dai colleghi dell'opposizione, a nome, credo, di tutto il centro-sinistra. Preciso subito che non intendo occuparmi di profili che abbiamo già affrontato discutendo la necessità e l'urgenza e che pure sono emersi nelle esposizioni dei colleghi. Non mi occuperò di qualche questione - mi perdonino i colleghi - minore, come la citazione del CNEL da parte del collega Eufemi, per carità, rispettiamo tutti, ma che sappiamo anche che da tanti è ritenuto inutile, ancorché di rilievo costituzionale. Quindi, non è serio identificare nel merito una violazione di rilievo significativo della Costituzione.

una disciplina saldamente radicata nella potestà legislativa dello Stato. La concorrenza, il mercato, i diritti dei consumatori e degli utenti fanno parte, al di là di ogni ragionevole dubbio, della potestà esclusiva - tra l'altro - dello Stato. Ci possono essere singoli profili di rapporto con materie che hanno anche connotazioni di competenza concorrente; la Camera ha inoltre introdotto taluni punti di richiamo della potestà regionale, ma nel suo complesso la materia si lega per la funzionalità a interessi che sono con certezza riferiti alla potestà legislativa dello Stato. Poi c'è un complesso di argomenti che ha a che fare con quello che uno dei colleghi ha definito il ritorno ai prezzi amministrati. Mi riferisco al problema della ricarica dei telefonini al fatto che si sia andati a incidere su tematiche di mercato. In merito,

ancorché autorevoli, ma minoritarie, nel senso che esso abbia una tutela implicita; nessuno dubita che ci siano però interessi generali e sociali prevalenti sul mercato ai sensi della Costituzione. In ogni caso, vorrei segnalare ai colleghi che hanno prospettato questo tema che nessuno sta riportando in vita un sistema di prezzi amministrati. Qui il problema è altro. La domanda è: può il legislatore, soggetto politicamente responsabile, intervenire per eliminare anomalie del mercato, puntuali e specifiche, comportate dal fatto che solo in questo Paese esistono alcuni particolari balzelli? È vero che c'è un'autorità nel caso dei telefonini; l'autorità avrebbe potuto intervenire, sicuro, ma non lo ha fatto: ha in realtà impiantato una procedura che è durata mesi. Il Governo ha ritenuto di intervenire con un proprio

un'attività speculativa da parte dei gestori della telefonia. Qui ognuno deve fare il suo mestiere. L'autorità probabilmente non lo ha fatto prima, quando poteva e doveva; il legislatore si è riappropriato del tema e l'autorità, come può e deve, lo faccia adesso. Il collega Pastore ha sottolineato un punto di particolare delicatezza, quello della revoca, richiamando una storia normativa.

collega Pastore, se è una scelta di civiltà che alla revoca si accompagni il lucro cessante al danno emergente. La domanda, in termini costituzionalistici, è un'altra e può essere semmai questa: si giustifica una asimmetria, nel caso della revoca, per cui il risarcimento si ha soltanto per il danno emergente e non per il lucro cessante? Questo è il

La revoca non significa che la pubblica amministrazione si alza la mattina e cambia idea, perché così le aggrada, ma vuol dire che c'è un interesse pubblico prevalente e preminente che giustifica il capovolgimento di una decisione già assunta. porre la questione in questi termini: l'esistenza di un interesse pubblico prevalente e preminente giustifica o no la asimmetria nella disciplina? Giustifica che si abbia la revoca senza danno? Il recupero del danno emergente significa infatti che comunque il privato non riceve danno; quello che non consegue è il lucro sperato, il profitto che avrebbe dovuto avere. Non voglio fare questioni filosofiche. Chiedo tuttavia se veramente pensiamo che non sia tollerabile, in termini costituzionali, che in presenza di un interesse pubblico preminente il privato veda il ristoro soltanto del danno che subisce e non del profitto che perde. Mi permetto di dubitarne. Si può discutere se ciò sia opportuno o meno; ma la costituzionalità è un'altra cosa. Si suggerisce inoltre che vi siano interessi occulti, per cui si è cambiato; queste sono illazioni che respingo, e che comunque non hanno niente a che fare con la Costituzione. Il collega Grillo afferma che non si può intervenire sull'autonomia privata. Collega Grillo, è puramente falso. Se così fosse, noi non potremmo fare una legge sull'equo canone; ma nessuno ritiene che ciò non possa essere fatto. È la stessa cosa, tale e quale;

(è esattamente quello che dicevo prima). La Costituzione vigente (forse non quella che il collega Grillo vorrebbe vigente) consente alla preminenza di interessi di altro genere, in particolare di interessi sociali, su valori che pure hanno un rilievo costituzionale, ma che non sono che non sono parificati. Noi non potremmo, se fosse vero l'assunto del collega Grillo, costringere le società assicuratrici a mollare la presa con la quale hanno azzannato i poveri assicurati in questo Paese e, in qualche caso, li hanno dissanguati. È il caso, ad esempio, della responsabilità civile, per cui le società assicuratrici sono state condannate (purtroppo invano) ad una megamulta dall'Autorità per la concorrenza e per il mercato (cioè quel valore che il collega Grillo giustamente Capisco, signor Presidente, che si vogliano difendere in quest'Aula interessi assai corposi. È una cosa legittima, è una scelta che fa parte della politica; ma non facciamo finta che abbia a che fare con la Costituzione. Non diciamo quindi che siamo di fronte ad un'usurpazione della legalità da parte dal legislatore. Io dico che noi oggi vediamo il recupero di un interesse pubblico di cui si era fatto strame da parte del precedente Governo. *(Applausi dal

Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che ci accingiamo a discutere e approvare, si inserisce nell'ambito di un percorso di politiche di tutela del consumatore e di liberalizzazione più ampio, avviato dal Governo con il decreto-legge del luglio scorso, e proseguito successivamente con numerosi altri provvedimenti che, nel loro insieme, hanno inteso perseguire l'obiettivo di un più ampio sviluppo dell'economia e di un più efficiente funzionamento dei servizi offerti al cittadino. Risulta incomprensibile l'atteggiamento ostruzionistico, tenuto in particolare alla Camera dei deputati, dalle forze del centro‑destra, che mentre propugnano a parole il liberismo, la concorrenza e le tutele, nei fatti, quando erano al Governo, nulla hanno fatto per avviare politiche di liberalizzazione e di tutela del consumatore. È quindi logico forse, per coprire il loro fallimento, che nel corso del dibattito svoltosi nei giorni scorsi alla Camera abbiano tenuto di fatto un comportamento ostruzionistico, per cercare di impedire la conversione del decreto. E qui al Senato, paradossalmente, i colleghi della Casa delle Libertà si lamentano per la ristrettezza dei tempi di discussione a cui siamo costretti dal comportamento dei loro stessi colleghi di partito. deputati la maggioranza ha svolto un lavoro di confronto e di approfondimento prima con le associazioni di rappresentanza e, successivamente, ha aperto un dialogo reale all'interno della competente Commissione e della stessa Assemblea. Non si può quindi parlare di una maggioranza chiusa su se stessa, quando dal confronto sono state accettate ben 36 modifiche, di cui 21 proposte dalla minoranza. La posizione del centro‑destra, che da una parte parla di un provvedimento che non ha contenuti e dall'altra tenta in ogni modo di ostacolarne l'approvazione, mi appare come una tattica di difesa dei particolarismi e dei corporativismi contro l'interesse delle famiglie italiane, che da questo provvedimento potranno risparmiare alcune centinaia di euro all'anno, che non sono poca cosa per chi magari ha un reddito attorno ai 1.000-1.200 euro Il decreto-legge che abbiamo oggi alla nostra attenzione si inserisce nel tracciato disegnato dai precedenti provvedimenti e prosegue nell'azione di rimozione degli ostacoli posti da norme protezionistiche a tutela degli interessi di pochi, da procedimenti inutilmente complessi e farraginosi che rallentano lo sviluppo economico e imprenditoriale. Introduce invece norme che rendono più concorrenziali gli assetti del mercato, favoriscono la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei princìpi comunitari in materia e garantendo una maggiore tutela del cittadino. Con il decreto-legge n. 223 del luglio 2006, il Governo ha voluto dare un primo forte segnale al Paese sulla strada delle liberalizzazioni in taluni settori produttivi e professionali; gli interventi normativi ivi previsti, alcuni dei quali raccoglievano segnalazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stati accolti positivamente dall'opinione pubblica e ora, a distanza di alcuni mesi dalla loro approvazione, iniziano a produrre i risultati attesi. In breve, le misure sulla liberalizzazione della vendita dei medicinali da banco hanno consentito l'apertura su tutto il territorio nazionale di circa un migliaio di nuovi esercizi tra farmacie e parafarmacie, di cui circa il 15 per cento all'interno della grande distribuzione, nonché un abbattimento dei prezzi di vendita dei farmaci, in media del 20 per cento, spinti verso il basso dai prezzi praticati dai nuovi esercizi. Le disposizioni sul potenziamento dei servizi di taxi iniziano a produrre i primi risultati positivi ed in parte inattesi, stante la forte protesta iniziale e gli scioperi proclamati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei tassisti. Le disposizioni sui passaggi di proprietà delle autovetture, con l'abolizione del ricorso obbligatorio al notaio, hanno consentito un notevole abbattimento dei costi legati a tali operazioni e uno snellimento dei tempi e delle procedure amministrative, che nell'85 per cento dei casi vengono ora svolte da agenzie di servizi automobilistici. Sempre in ambito assicurativo, a pochi mesi dall'avvio, si segnala l'affermazione e il gradimento che sta ottenendo il risarcimento diretto dei sinistri da parte delle assicurazioni. Le misure relative all'eliminazione dei costi di chiusura dei conti correnti bancari, inizialmente contrastate dal mondo bancario, sono diventate ora un elemento di *marketing* pubblicitario delle banche, che ha portato ad un evidente abbattimento dei costi di gestione dei medesimi. Questi interventi, seppure parziali, hanno fornito una prima risposta alle esigenze manifestate da ampi settori della società e dell'economia italiana, che chiedevano al Governo atti concreti, da un lato contro le pratiche anticoncorrenziali determinate dalla difesa di interessi particolari e corporativi, e dall'altro a favore del libero accesso al lavoro e al mercato produttivo. Quindi, una risposta ai giovani ed a tutti coloro che intendono avviare nuove attività professionali ed imprenditoriali. A quel primo provvedimento, il Governo ha fatto seguire altre misure per l'allargamento della concorrenza dei mercati produttivi che, annunciate già nel DPEF 2007-2011, sono state successivamente introdotte nella finanziaria 2007 ed in altri provvedimenti di politica di liberalizzazione dei mercati, presentati all'esame del Parlamento. Tra questi segnalo: il disegno di legge delega per il completamento della liberalizzazione nei settori dell'energia e del gas naturale e per il risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; il disegno di legge delega per il riordino dei servizi pubblici locali; quello per l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori; il disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali; quello per il riassetto delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati; da ultimo il disegno di legge recante misure per il cittadino-consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali. Il provvedimento oggi in discussione prevede una serie di norme con cui il Governo si propone di rimuovere e rendere più trasparenti i comportamenti adottati dai gestori della telefonia mobile, di Internet e delle televisioni, dalle autostrade, dalle banche, dalle assicurazioni e dalle compagnie aeree, che hanno avuto come conseguenza costi aggiuntivi e ingiustificati per i consumatori, che invece, grazie al decreto che stiamo convertendo, saranno rimossi. Desidero mettere in rilievo solo alcuni aspetti per me più significativi di questo provvedimento. Viene disposta la soppressione dei costi di ricarica dei cellulari e dei servizi Internet e *pay* TV, finora richieste dai gestori e che rappresentano un costo aggiuntivo rispetto al costo del traffico richiesto; è una tassa ingiusta che prescinde dal servizio utilizzato. Si prevedono misure per una maggiore informazione degli utenti della rete autostradale, in relazione ai prezzi del carburante e al traffico sulla rete; si interviene per disciplinare il fenomeno della pubblicità, a volte ingannevole, sulle tariffe per il trasporto aereo per i passeggeri; si dispone che l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale o allo svolgimento di attività economica o professionale non deve essere in nessun caso onerosa per il debitore, mentre, per i mutui già stipulati che prevedono da contratto oneri a carico del debitore, in caso di estinzione anticipata, è prevista una fase di rinegoziazione tra l'ABI e le associazioni dei consumatori; si introduce inoltre la portabilità del mutuo da un istituto di credito all'altro senza oneri aggiuntivi. Vengono poi introdotte disposizioni per incrementare la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore assicurativo; si introduce il divieto di addebitare, nei rapporti assicurativi e bancari, al cliente le spese di predisposizione, produzione e spedizione. Oltre a queste misure che più direttamente fanno riferimento alla convenienza per i cittadini, si semplificano le procedure di avvio e di cessazione delle attività imprenditoriali, introducendo la comunicazione unica: l'imprenditore con una semplice comunicazione inviata, anche per via telematica o su supporto informatico, all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, elimina una serie di adempimenti amministrativi finora previsti, quali l'iscrizione al registro delle imprese, all'INPS, all'INAIL, nonché le pratiche atte all'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Con la presentazione della comunicazione unica l'imprenditore ottiene dallo sportello della camera di commercio una ricevuta che gli consentirà l'avvio immediato dell'attività imprenditoriale ed entro sette giorni dovrà ottenere i dati definitivi dalle amministrazioni competenti. Si prevedono inoltre apposite misure per facilitare l'accesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e professionale di acconciatore, estetista, pulizia e disinfezione, facchinaggio, autoscuole e guide turistiche. Anche in questo caso sarà sufficiente la sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del Comune. Decadono conseguentemente tutti i vincoli relativi alle distanze minime tra esercizi, al numero massimo dei soggetti che svolgono la medesima attività e al rispetto dell'obbligo di chiusura settimanale. Questo consentirà una maggiore espansione di tale attività, con riflessi positivi sull'occupazione, e creerà maggiore concorrenza e, quindi, una migliore qualità dei servizi. Si garantisce inoltre ai giovani un sistema di formazione scolastica, più legato al mondo del lavoro, adeguato e paragonabile a quello del resto dei Paesi comunitari, che consenta loro di rispondere alle nuove esigenze di preparazione professionale provenienti dal mercato del lavoro. Per concludere, tralasciando altri aspetti importanti solo per ragioni di tempo, voglio ricordare che, al fine di consentire la realizzazione del sistema di alta velocità sulle tratte indicate nel decreto, nel rispetto delle norme europee, si prevede la revoca delle concessioni rilasciate da precedenti Governi - si parla di circa sedici anni fa - in deroga a tale normativa dall'Ente ferroviario di Stato alla TAV per la realizzazione di alcune tratte ferroviarie. I lavori verranno affidati con gare ad evidenza pubblica, ristabilendo i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa; risparmiando risorse pubbliche, dal momento che i costi di quei progetti sono lievitati del 400 per cento; prevedendo forme di rimborso per le spese di progettazione sostenute dai *general contractor.* E' questo - a mio avviso - l'unico modo per dar finalmente corso a quelle opere. Per i motivi sopra esposti, ritengo che bene facciamo a voler convertire il decreto in legge perché il Paese aspetta questo provvedimento, che sicuramente avvantaggerà il Paese stesso e i cittadini, che ne trarranno benefici sia economici, sia in termini di qualità dei servizi.

osservo i provvedimenti del ministro Bersani con lo stesso sguardo con cui Laocoonte guardava il cavallo di Troia: un involucro appetibile dal contenuto letale. Laocoonte, oggi, non viene strangolato da una serpe inviata da Poseidone, ma dalla minaccia del ricorso al voto di fiducia, che impedisce, in primo luogo, di dire al Paese la verità. Che si tratti di un progresso, è del tutto discutibile. Ma parlavamo di cavalli di Troia. Dunque, la prima lenzuolata Bersani ricopriva le vergogne del vice ministro Visco e, con le sue norme fiscali, puntava ad essere il sudario di tutte le migliaia di partite IVA non in grado di rivolgersi a costosi studi di commercialista. Oggi, la seconda lenzuolata vuole rappresentare il sudario su due provvedimenti essenziali: la riforma della scuola promossa dal ministro Moratti e la TAV, che, se venisse approvato il decreto, verrebbe rinviata al tempo del mai. Non solo, ma il solo proporre di stracciare patti sottoscritti con una regola in vigore dal 1991 - è bene ricordarlo - rappresenta la campana a morto nei confronti di investitori da attrarre sul terreno essenziale delle infrastrutture. E con che soldi vogliamo fare le infrastrutture? O, nonostante l'impegno, che volentieri riconosco, del ministro Di Pietro, l'obiettivo di una parte della maggioranza sarebbe quello di ridurci all'uso del calesse? Così, per decreto, con voto di fiducia, senza che il Parlamento abbia la possibilità di svolgere la propria funzione, che non può essere limitata alla ginnastica che tutti noi compiamo schiacciando un bottone, si cerca di mettere la parola fine a un'opera essenziale, ignorando gli sguardi sbalorditi dei nostri *partner* europei. Questo provvedimento rappresenta, innanzitutto, più che una liberalizzazione, una museruola inaccettabile, che dovrebbe essere rifiutata prima di tutto da coloro che si sciacquano la bocca con la parola democrazia. Una museruola che strangola il dibattito parlamentare, una lenzuolata che copre, anche su questo terreno, le irriducibili divergenze politiche della maggioranza numerica che sorregge il Governo Prodi. Che forse può decidere, approfittando dell'ipocrisia di alcuni, ma non può discutere, correndo il rischio di dividersi. Già il dibattito alla Camera ha posto in luce come la seconda lenzuolata utilizzi impropriamente il termine «liberalizzazioni» e il termine «modernizzazioni». Vale la pena riprendere per sommi capi che per liberalizzazioni e modernizzazioni si spacciano l'abolizione delle ricariche, che verrà ricaricata sulle tariffe, l'abolizione della penale sui mutui, che verrà ricaricata sugli interessi e che del resto già faceva parte delle offerte di alcune banche, la beffa di adempimenti burocratici per la costituzione di un'impresa che vengono posticipati anziché essere aboliti. Le sue liberalizzazioni, ministro Bersani, sono una merce contraffatta, che solo un'accorta campagna di stampa è riuscita a mascherare. In un Paese dalla civiltà giornalistica migliore della nostra, lei sarebbe stato messo in difficoltà, nonostante i suoi modi concreti e simpatici da emiliano verace. Non si parla della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che resta bloccata in quest'Aula per insanabili dissidi all'interno della maggioranza. Non si parla di liberalizzazioni nei settori dei trasporti, dell'energia, delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e delle tariffe idriche. Insomma, ministro Bersani, avrebbe fatto meglio a rubricare questo testo sotto un altro titolo, poetico ma reale: «Questo solo possiamo dirvi, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».

Claudio Gentili, responsabile dell'area *educational* di Confindustria, proprio qualche giorno fa, esprimeva un aperto apprezzamento dell'articolo 13 del decreto oggi in discussione.

congruità di questo decreto anche in materie che sembrerebbero estranee all'obiettivo prioritario, cioè lo sviluppo economico, l'innovazione del sistema Paese), su quel famoso articolo 13, che, con un grande e ricco lavoro dei nostri colleghi alla Camera,

Claudio Gentili scriveva che le industrie nel nostro Paese cercano ogni anno 550.000 profili di alta professionalità tecnica e non li trovano. cuore dell'articolo 13 di questo decreto, che tratta temi anche più importanti della professionalità tecnica - quali il tentativo di superare la mortalità scolastica, la dispersione degli istituti professionali, non dei tecnici, dei corsi triennali delle Regioni, non dei corsi triennali degli istituti professionali di Stato (quindi c'è una parte del decreto che affronta questioni ancora più dense, più prioritarie, che attengono alla cittadinanza, ai diritti di istruzione) -

mettere in moto un volano effettivo per lo sviluppo economico del Paese. Il giudizio del responsabile dell'area *educational* di Confindustria, giudizio neutro,

delle possibili elargizioni liberali deducibili o detraibili di singoli cittadini, associazioni, famiglie, enti economici e imprese, con garanzie di non governare la giunta esecutiva dell'istituto, naturalmente, che nella relazione tecnica viene calcolato approssimativamente al 33 per cento dell'attuale somma delle erogazioni liberali. Vuol dire ogni anno 140 milioni di euro.

cultura solidaristica e liberale insieme. Il terzo punto così importante dell'articolo 13 è la sollecitazione forte, attraverso il *master plan* individuato tra Governo e sistema delle autonomie locali, all'attuazione degli articoli 117 e 116 della Costituzione, vale a dire alla riforma federalista del sistema dell'istruzione professionale, che paradossalmente è compatibile con l'assunzione forte del peso della formazione tecnica nel sistema statale di istruzione. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nella nostra discussione

che riemerge periodicamente, del ruolo del Senato, o meglio di questa Camera, su questo specifico provvedimento, così come è accaduto alla Camera in precedenza per altri provvedimenti. Si

più che concentrarsi sul merito del provvedimento, si sofferma su altro, per cui altre cose prevalgono nella discussione. L'ostruzionismo praticato alla Camera rientra sicuramente in pieno - lo abbiamo praticato anche noi nella scorsa legislatura nella disponibilità dei colleghi del centro-destra di valutare la propria azione, ma anche la difesa della validità del decreto-legge in esame, e quindi della nostra strenua opposizione alla sua decadenza, è assolutamente una nostra legittima prerogativa, dunque una prerogativa della maggioranza. E qui, tra questa contesa, si è sviluppata la discussione. Ritengo che la scelta

Ora, perché si è scelta da parte dei colleghi del centro-destra questa linea? Perché si è enfatizzato il significato di alcune norme tanto da porre in essere una pratica ostruzionistica, sempre legittima salvo non diventi un costume abituale nella condotta dei nostri lavori parlamentari? L'eccezionalità del contenuto non sembra giustificare tale atteggiamento, né tanta ostilità e tanta ostilità e tanta opposizione. La risposta forse va ricercata in una valutazione politica, che ancora una volta si è rivelata sbagliata. Come Come avete sbagliato l'altro ieri sull'Afghanistan per il rifìnanziamento della missione militare italiana, continuate a sbagliare anche su questo provvedimento, rifiutando di misurare l'iniziativa politica in proporzione al merito delle questioni di cui si discute. il provvedimento affronta una serie di questioni sulla linea di quanto già fatto con il decreto dello scorso luglio. Come sappiamo, l'Italia è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei nell'apertura del mercato interno ad una piena e concreta competizione per le merci ed i servizi. Esiste ancora una serie di lacci ed impedimenti gravanti sul sistema economico ed amministrativo autorizzativo, accompagnati da balzelli e costi impropri a carico dei consumatori. L'accesso alle attività professionali e libere non è libero come dovrebbe essere. In altri termini, non si compete virtuosamente e inoltre si scaricano sul consumatore - anello tradizionalmente più debole della catena costi impropri sui medesimi beni e servizi assenti negli altri Paesi europei. Mi chiedo il motivo per cui fra noi non ci sia accordo sul fatto che non è giustificato pagare la ricarica dei telefonini, contrariamente a come accade nel resto d'Europa, pagare una penalità se si decide di estinguere anticipatamente un mutuo per la casa

in un Paese normale come dovrebbe essere il nostro, non ci troviamo d'accordo e invece questo dibattito mette in evidenza che siamo gli uni contro gli altri. Si tratta di un'anomalia che noi vorremmo

è diverso l'atteggiamento che avete quando si discute di questioni concrete. Tremonti alla Camera ha persino rispolverato la *perestroika* sovietica per giustificare la sua posizione di ostilità.

le cose vanno meglio di come andavano durante il Governo di centro-destra. L'economia si è rimessa in moto, non siamo più, almeno per ora, il fanalino di coda nella crescita dell'Europa e persino nel rapporto con il fisco il sistema italiano mostra tendenze alla normalità; in altri termini, si evade e si elude meno di prima, così si determina per il combinato effetto di questi due fattori una crescita del gettito fiscale. Le misure previste in finanziaria in questo quadro cominciano ad apparire più eque di quanto la passata discussione non sia riuscita ad evidenziare, i conti sono più in equilibrio e si riguadagna terreno

in cui rilanciare più efficacemente le riforme e l'apertura del sistema alle liberalizzazioni; dovremmo discutere di più di ciò che fanno ENI, ENEL e così via. Signor Ministro, sarebbe opportuno che potessimo discutere anche in questa sede, visto che siamo i principali azionisti e deteniamo le quote di maggioranza relativa,

di soli emendamenti soppressivi, nella sostanza non produciamo emendamenti migliorativi e che rilancino in questa direzione. In conclusione, signor Presidente, a nostro avviso occorre scegliere questo terreno: la nostra disputa - se vi sarà - verrà vissuta come un confronto per migliorare e creare condizioni di crescita del nostro sistema economico, non per impedire al Governo di operare e alla sua maggioranza di esistere. Dopo dieci mesi di attività piena, siamo ancora alla ricerca di un possibile confronto con i liberali del nostro sistema politico presenti nel centro-destra: si decidano a battere finalmente un colpo. Signor Presidente, colleghi senatori, siamo chiamati, ancora una volta, ad esprimerci,

Siamo, ormai, al paradosso: nella storia del Parlamento non è mai avvenuto che un decreto-legge arrivasse al Senato negli ultimi cinque giorni utili per la sua

Si è anche detto che tale urgenza derivi dalla necessità di approvare il provvedimento prima della scadenza del sessantesimo giorno di ragionare, cari colleghi, sul fatto che più di due settimane sono state perse dall'Esecutivo - e dalla maggioranza che lo sostiene - per verificare la propria tenuta, fare la conta dei voti disponibili e correre ai ripari per la crisi di Governo.

non aumenta la concorrenza, anzi, in alcuni casi ne riduce la possibilità; non apporta migliorie né risparmi alla pubblica amministrazione; può ingenerare disservizi, minore tutela e maggiori costi per i cittadini. Cominciamo dalla prima misura inserita nel testo, sicuramente di maggior effetto e grande impatto giornalistico e mediatico, in quanto azzera i costi di ricarica telefonici. Se ci

La stessa Unione Europea, nei giorni scorsi, ha espresso perplessità circa gli effetti reali di tale misura. Ugualmente di scarso effetto appare la misura relativa alla liberalizzazione del sistema della distribuzione della benzina nel nostro Paese. Se scendiamo poco sotto la superficie del ragionamento, ci rendiamo conto di come l'effetto sui consumatori sia estremamente minimale. Il prezzo della benzina, infatti, non può certo dipendere dal singolo benzinaio, in quanto è necessariamente legato alle problematiche di carattere internazionale (e, soprattutto, alle politiche messe in campo dalle compagnie petrolifere, che realizzano cartelli a danno dei consumatori), non certo ai singoli distributori. Ciò nonostante, si è preferito scegliere il bersaglio più facile, colpendo i benzinai, invece di sanzionare o, comunque, regolare meglio le compagnie petrolifere. Vale la pena soffermarsi anche sulla norma che dovrebbe permettere la creazione di un'impresa in un giorno, come recita quello che sembra più uno *slogan* che il titolo di un articolo disegno Al riguardo, infatti, resta da vedere quali saranno i Regolamenti attuativi, per capire se davvero sarà possibile far nascere in Italia un'impresa in un giorno (specialmente a fronte di una macchina burocratica che resta estremamente pesante

Il resto del decreto prevede tutta una serie di interventi che, più che liberalizzazioni, appaiono misure sui prezzi (come l'eliminazione di vincoli e la velocizzazione delle procedure per aprire attività imprenditoriali). Si tratta, in sostanza, di un decreto contenitore con dentro di tutto un po', a mio avviso troppo ampio ed eterogeneo per essere veramente utile ed efficace. Non regge, al riguardo, neppure la favola che vuole che l'urgenza di trattare tali argomenti insieme e contemporaneamente sia dettata dalla necessità di agganciare il treno della ripresa economica che è in atto e favorirla con nuovi provvedimenti. La crescita economica del nostro Paese non è certo stata accelerata dal DPEF approvato dal Governo Prodi, dall'ultima legge finanziaria, né, tantomeno, dalle recenti misure sulle liberalizzazioni del precedente decreto Bersani-Visco dello scorso autunno. hanno appesantito, semmai, di nuove tasse e balzelli. Al riguardo, non farebbe male un po' di onestà intellettuale nel considerare che l'andamento dell'economia di un grande Paese come il nostro è inevitabilmente legato ad una serie di variabili indipendenti, quali gli accadimenti internazionali, gli andamenti dell'economia globale, oltre che l'azione dei Governi, i cui effetti si dispiegano ed affondano le loro radici in periodi sicuramente più lunghi di un paio di anni. Come detto, e mi avvio a concludere, in questa nuova legge c'è un po' di tutto: dai provvedimenti sulle ricariche telefoniche agli interventi sul rimborso delle assicurazioni, a quelli sul reintegro dei mutui, sino alle procedure per iniziare un'attività imprenditoriale, all'eliminazione dei vincoli sulle professioni di panificatori, estetisti, acconciatori, guide turistiche per finire con le licenze delle autoscuole. Resta da vedere se poi queste misure calate dall'alto, senza neppure un briciolo di concertazione con le parti interessate, potranno davvero sortire gli effetti sperati. Mi viene da chiedere se davvero l'*Authority* sulle telecomunicazioni sarà in grado, con gli attuali strumenti, di arginare l'attività delle società telefoniche sicuramente già attivatesi per studiare nuovi modi per recuperare i mancati introiti sui costi di ricarica. Pur volendo sorvolare sul contenuto dei primi articoli, non può passare sotto silenzio il fatto di aver inserito un pezzo di riforma della scuola in un decreto-legge fatto passare con la fiducia alla Camera e al Senato. Appare francamente inaccettabile, non solo nel merito, ma anche nel metodo, la volontà di intervenire pesantemente sul testo della riforma Moratti, in una materia delicata come quella della scuola, senza avviare un briciolo di confronto o dibattito nel Paese ed in Parlamento, preferendo smontare l'impianto della legge pezzo su pezzo, con decisioni parziali o decreti, com'è stato fatto con l'abolizione della sperimentazione, poi con l'abolizione della figura del *tutor*, adesso con l'abolizione del liceo economico e tecnologico

(come al Senato) è stata affrontata nella Commissione attività produttive, che trova la sua ragione d'essere nel fatto che questa maggioranza non ha la forza di affrontare un dibattito parlamentare su temi di grande importanza ed è costretta ad *escamotage* tecnici e forzature per tirare avanti e sopravvivere sulle spalle degli italiani, che meriterebbero un Governo ed una guida in grado di assumere decisioni e con la forza di sostenerle in sede parlamentare, senza ogni volta dover passare sotto le forche caudine di questo o quel partito, di questo o quel senatore, che potrebbe compromettere l'esito della votazione. In conclusione, si tratta di un provvedimento, per la maggior parte del suo contenuto, di scarsa efficacia, più di propaganda che di sostanza. L'impressione che lascia è quella di un'ennesima occasione persa sul piano delle liberalizzazioni e di un'occasione carpita al volo per cancellare subdolamente un altro pezzo della riforma del Paese avviata dal Governo Berlusconi.

un mercato più aperto in cui si riducano le rendite di posizione, capace di riconoscere i diritti dei consumatori è un fattore determinante per lo sviluppo e la crescita. Tale è il messaggio chiaro che con questo decreto vogliamo dare al Paese. Proprio questo terreno di iniziativa, che una certa semplificazione definisce liberalizzazione, ci consente di trovare una nuova sintesi tra diritti finora inesplorati e crescita economica. Sono tante le spese che questo decreto permette di ridurre, aumentando la concorrenza e senza costi per il bilancio pubblico. È evidente come eliminare oboli impropri, come le ricariche telefoniche, oppure garantire una maggior concorrenza sui mutui restituisca risorse ai cittadini. È altrettanto evidente che, in proporzione al reddito, sono proprio le fasce più deboli a ricevere un maggior vantaggio da questa restituzione. Facciamo queste scelte con la consapevolezza che un mercato distorto può forse garantire qualche rendita di breve periodo, ma non consente al Paese di essere competitivo di fronte alle sfide internazionali. Ecco come con questo provvedimento noi riusciremo a coniugare equità e sviluppo. Il punto allora non è quello di difendere chi, impaurito dal cambiamento, si batte per mantenere vere e proprie incrostazioni, ma semmai fare di più, agire con maggiore convinzione e radicalità. Si pensi, ad esempio, al grande tema dell'accesso alle professioni liberali. Se vogliamo rafforzare la crescita, di cui vediamo ora i primi segnali, garantire al nostro Paese uno sviluppo solido e assicurare la coesione sociale, serve coraggio sulla strada tracciata da questo provvedimento e da quelli che lo hanno preceduto. Ma serve anche la consapevolezza delle priorità. Per rafforzare lo sviluppo delle attività economiche, una delle finalità di questo decreto, il ruolo della scuola e dell'istruzione tecnica e professionale è centrale. centrale. Valorizzare l'istruzione tecnica e professionale consente di ridare slancio alle nostre imprese e al nostro tessuto produttivo. Se vogliamo uno sviluppo duraturo e non effimero dobbiamo affidarci all'istruzione. Ci sono stati, nella storia del nostro Paese, alcuni modelli che hanno fondato la propria crescita su elementi diversi dalle competenze; basti pensare al tanto decantato modello Nord-Est, una delle aree del Paese che negli anni '90 aveva, allo stesso tempo, uno dei tassi di crescita più significativi e uno dei tassi di abbandono scolastico più alto. Tocchiamo ora con mano le conseguenze di quel modello: appena l'ingresso dei Paesi dell'Est nell'Europa ha consentito di accedere a manodopera a basso costo, tanti di quei ragazzi che avevano abbandonato la scuola per soddisfare il proprio desiderio di consumi e autonomia si sono ritrovati espulsi dal mercato del lavoro. Esiste invece un altro esempio, quello del *boom* degli anni '60, in cui la scuola media unica e obbligatoria, introdotta nel 1962, e un sistema di istruzione tecnica e professionale di eccellenza hanno avuto un ruolo rilevantissimo. Si pensi ai periti chimici, che hanno sostenuto la nascita della chimica italiana, o ai periti industriali o elettronici. La ricchezza di quegli anni ha camminato anche sulle gambe di quei lavoratori specializzati. Oggi, con gli interventi di riforma profondi che si introducono con questo decreto abbiamo l'ambizione di riavviare quel percorso di ricchezza e di crescita. Questa è la nostra ambizione, che passa necessariamente per la via del superamento del cosiddetto progetto Moratti. Il superamento del modello duale e l'eliminazione dei licei tecnologico ed economico consentono di rilanciare quell'istruzione tecnica e professionale che sono state per anni una vera e propria eccellenza nel panorama della scuola italiana ed europea. Questo rilancio consente anche di rendere più chiara la dizione poco puntuale introdotta nel 2001 nel Titolo V della Costituzione: l'istruzione professionale torna ad essere un pezzo del sistema di istruzione secondaria, competenza esclusiva dello Stato. In questo contesto, assicurare all'istruzione professionale la continuità della sua funzione rispetto agli attestati di qualifica sarebbe un ulteriore elemento di chiarezza. E' evidente come questi elementi saranno maggiormente chiari quando cominceremo a vedere i frutti della scelta dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni. Mancando ancora una esperienza consolidata sul campo, oggi risulta più difficile cogliere i diversi momenti di integrazione tra i vari sistemi. Ma questo non può essere un alibi ad alcune scelte

se non si ha un generale incremento delle competenze teoriche, culturali, linguistiche. L'altro elemento alla nostra valutazione è quello relativo alle detrazioni e deduzioni per il sostegno che le famiglie e le imprese vogliono mettere a disposizione delle scuole. Il ruolo delle imprese, in particolare, è un elemento delicato. Non abbiamo difficoltà a sostenere la soluzione delle deduzioni, visto che ancora non siamo di fronte all'ingresso delle rappresentanza delle imprese nel consiglio di istituto. È evidente, però, come sia difficile una discussione in due tempi, sul decreto da un lato e sul disegno di legge sulle liberalizzazioni dall'altro. In quella sede, coerentemente con il sostegno che diamo oggi sulle deduzioni, saremo rigorosi nell'affermare la centralità, negli organi collegiali, di chi vive e lavora nelle scuole, cioè studenti, famiglie e insegnanti. Così come questa scelta dei due tempi tra le proposte normative rende difficile la discussione sul fondo perequativo, che è necessario se si introducono le detrazioni e che avremmo preferito vedere in questo testo. La scuola sta già compiendo grandi sacrifici a causa delle scelte compiute in finanziaria e ridurre ulteriormente gli stanziamenti, in particolare quelli per l'elevamento dell'obbligo, soprattutto in assenza del fondo perequativo, è una scelta sbagliata. Restano alcune ombre: la prima è che il carico economico dovuto per le detrazioni sia a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione e non del Ministero dell'economia. Speriamo che l'ordine del giorno presentato su questo decreto possa consentire, nel medio periodo, di rivedere tale scelta. La seconda perplessità è che il bilancio dello Stato sia eroso dalle detrazioni donate alle scuole private. Noi per senso di responsabilità abbiamo accettato, con la finanziaria, un aumento di 100 milioni al fondo per le scuole non statali, nonostante una grande e radicata perplessità. Non si capisce perché, allora, le detrazioni per le donazioni alle scuole private non siano caricate su quel fondo, come sarebbe stato logico. Noi possiamo anche ammettere, visto che esiste la legge di parità, che le detrazioni vengano concesse anche per le private, ma se esiste una specifica unità previsionale nel bilancio è assolutamente irragionevole che non si usino quei soldi per la loro destinazione più logica. Nonostante quest'ultima perplessità, noi sosterremo la conversione del decreto, non per spirito di coalizione, ma perché facciamo una valutazione complessiva degli effetti benefici che le sue scelte hanno e avranno sulla vita dei cittadini. È altrettanto evidente, però, come sia urgente una più ampia e distesa discussione, in occasione del disegno di legge dovrà essere l'occasione per completare il disegno avviato con questo provvedimento con sempre maggior forza, coerenza, coraggio. Signor Presidente, onorevole ministro Bersani, avendo solo cinque minuti a mia disposizione limiterò il mio intervento alla questione della revoca delle concessioni TAV, la cui portata dirompente forse non è del tutto chiara a questo ramo del Parlamento. Voglio ricordare che con l'articolo 13 del testo in esame si intendono cancellare *tout court* le concessioni a suo tempo sottoscritte con i *general contractors* delle tratte ferroviarie Genova-Milano, Milano-Verona e Verona-Padova. Si tratta di un'iniziativa autolesionistica per il nostro Paese, perché di fatto sancisce il definitivo *de profundis* per la realizzazione del Corridoio ferroviario 5, che a questo punto escluderà l'Italia, ed è addirittura illegittima sul piano giuridico, con conseguenze gravissime per tutto l'ordinamento interno e di un *vulnus* inaccettabile nel corretto rapporto tra il pubblico e il privato. Come ha avuto modo di dichiarare un politico al di sopra di ogni sospetto l'onorevole Mantini della Margherita, che tra l'altro è anche un illustre docente di diritto amministrativo, la norma di cui stiamo discutendo può essere considerata un vero e proprio «esproprio stalinista e illiberale, che riporta la pubblica amministrazione in un'antistorica ed esagerata sfera di supremazia sul privato». Ripeto, sono queste le parole testuali usate da un autorevole esponente della maggioranza, che siede nell'altro ramo del Parlamento, per descrivere l'abominio giuridico che state avallando. Tutti i presupposti su cui si basa questo testo di legge sono documentalmente falsi e privi di ragionevolezza. È falso, infatti, che mettendo a gara le linee oggetto di revoca si possano realizzare dei risparmi finanziari, in quanto l'esperienza insegna che i ribassi d'asta sono dei risparmi illusori che generano successive richieste di adeguamento e contenzioso. Inoltre risulta evidente che Ferrovie dello Stato non ha alcun titolo per utilizzare gli elaborati progettuali oggi a disposizione, che evidentemente appartengono ai contraenti generali e la cui rinnovata predisposizione non potrà che generare oneri aggiuntivi. Ma voglio soffermarmi in particolare su quanto disposto dall'articolo 13, comma Questa norma interviene a modificare il testo dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Come è noto, quest'ultima norma sancisce il diritto ad un indennizzo a favore del privato, quando la pubblica amministrazione dispone la revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, ed è stata introdotta nel nostro ordinamento nella scorsa legislatura, a conclusione di un lavoro parlamentare *bipartisan* - ricordo a tale proposito che alla Camera il relatore del provvedimento fu all'epoca l'onorevole Bressa -, e costituiva il punto di arrivo di un faticoso percorso della dottrina e della giurisprudenza amministrativa sviluppatosi nell'arco di oltre un decennio. Ora il Governo intende scardinare tale principio generale di civiltà giuridica, introducendo proprio il comma 8-*duodevicies*, che prevede invece di ridurre ad un importo quasi simbolico l'indennizzo da corrispondere ai privati contraenti, che, anche senza colpa, vengono a subire la revoca di un contratto, e sottolineo di un contratto, liberamente sottoscritto con una pubblica amministrazione. C'è forse qualcuno in quest'Aula che crede che il diritto che si intende introdurre per la nostra pubblica amministrazione di calpestare la certezza del diritto acquisito con un contratto favorisca la credibilità dell'Italia agli occhi degli investitori esteri? Quindi, per spendere meno nella realizzazione delle linee ferroviarie (almeno è questa a parole la vostra intenzione, che peraltro resterà una pia illusione), nell'illusione di realizzare qualche economia negli appalti del treno veloce, decidete di scassare l'intero equilibrio giuridico dei rapporti pubblico-privato, un equilibrio faticosamente conseguito nel nostro ordinamento nel corso di decenni di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Avete la consapevolezza del mostro giuridico che state partorendo? Chi parla ha peraltro il fondato sospetto che la norma sia dettata dalla volontà di eludere surrettiziamente quanto è stato recentemente sancito negli arbitrati attivati dai *general contractors.* Voglio qui ricordare in particolare che un arbitrato promosso dal consorzio CEPAV DUE, *general contractor* per la tratta ferroviaria Milano-Verona, depositato in data 9 gennaio 2007, aveva già sancito la responsabilità di TAV Spa condannandola a corrispondere allo stesso consorzio il prezzo di tutte le progettazioni commissionate. Il giudizio è ancora in corso per l'ulteriore quantificazione del danno. In data 30 gennaio 2007, quindi proprio in corrispondenza dell'emanazione del decreto-legge che oggi stiamo discutendo, lo stesso consorzio ha introdotto un secondo arbitrato per l'accertamento dei danni subiti dal 2000 ad oggi. Se le cose stanno nei termini che ho denunciato, non possiamo dire che quella che state introducendo è a tutti gli effetti una norma *ad personam*, creata proprio per influire in un procedimento giudiziario in corso? A conclusione del mio intervento mi rivolgo al ministro Bersani, che sui *media* ha la pretesa di essere considerato un riformatore per eccellenza e non perde occasione di lanciare al centro-destra il guanto di sfida sulla capacità di essere autentici liberalizzatori. Signor Ministro, liberalizzare significa forse ridurre i costi di ricarica delle schede telefoniche, che i gestori di telefonia mobile stanno già recuperando attraverso una rimodulazione delle tariffe, perché altrimenti non sono in grado di far quadrare i loro conti, come lei fa oggi, o piuttosto essere liberalizzatori e liberali consiste nel contestare norme che introducono nell'ordinamento un "esproprio stalinista", per dirla con le parole dell'onorevole Mantini, come faccio io? E allora, ministro Bersani, provi a rispondere a questa domanda. In quest'Aula i veri liberali siamo noi o è lei? *(Applausi

e vedo che ciò sta avvenendo largamente anche nel dibattito. In un decreto sull'economia si compiono scelte importanti per la scuola. È uno scandalo? No, è un bene, un'opportunità, una forte scelta politica. È normale che sia così quando non si ha un senso residuale, da orto chiuso, dell'istruzione, ma un suo significato strategico: più scuola nell'economia, nella vita sociale del Paese, nel dibattito politico. Questa è la società della conoscenza, questa è l'economia basata sulla conoscenza. Nel decreto‑legge al nostro esame vi è appunto l'articolo 13, che reca disposizioni in materia di istruzione secondaria superiore e, in particolare, dell'istruzione tecnica e professionale, nonché agevolazioni fiscali per le donazioni a favore delle istituzioni scolastiche autonome, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa. Ecco, è un pensiero complessivo sul Paese: le cose necessarie, le cose urgenti, perché vi sia quel dinamismo che dalla vita economica e sociale alla vita, appunto, della conoscenza faccia decollare l'Italia. I primi mesi della legislatura - penso alla legge finanziaria, che contiene l'innalzamento dell'obbligo di istruzione - ci consegnano un approccio nuovo, che vede interventi sul sistema di istruzione con provvedimenti finalizzati allo sviluppo e al dinamismo economico del Paese. Il tema è chiaro. L'Italia sta affrontando una fase di cambiamento caratterizzata da interventi sulla struttura, sulla dinamica dell'economia e della crescita, sull'evoluzione sociale delle professioni e del Paese, sulla mobilità sociale, sul pieno utilizzo delle sue energie senza dispersioni; tutto ciò richiama quegli interventi sul sistema di istruzione che sono, a questo scopo, strategici. È il caso del rilancio della formazione tecnica e professionale, com'è della più efficace azione e programmazione delle attività delle istituzioni scolastiche attraverso il rafforzamento della gestione finanziaria, sostenuta dallo Stato, ma anche aperta al contributo del territorio. decreto noi abbiamo un rilancio, come non si era visto da molti anni, dell'area tecnico‑professionale nel sistema di istruzione del Paese. È il tempo nuovo dell'istruzione basata sulla crescita, che è la base della crescita. Ne è prevista l'urgenza, perché urgente è il rilancio del Paese. Proprio sul tema dell'istruzione tecnico-professionale vi sono i più recenti documenti della Commissione europea per una maggiore cooperazione, in Europa, in materia di istruzione e formazione tecnico-professionale, rendendo riconoscibili i crediti acquisiti nei diversi Paesi e le conoscenze professionali lungo l'arco della vita. E così, la stessa Europa consiglia un'ampia strategia che, tra i diversi obiettivi, pone l'accento sulle agevolazioni fiscali, che considera uno strumento politico potenzialmente importante per l'innalzamento del livello medio di capacità della popolazione, riconoscendo l'autonomia attribuita ai singoli istituti nel decidere contenuti, nell'assumere decisioni e nella destinazione dei fondi, per migliorare il rendimento degli studenti. È dunque il processo reale in atto, in Europa e in Italia, che consente di affrontare simultaneamente l'economia e l'istruzione e la formazione. Voglio notare che il contesto italiano ha visto in questi anni diminuire fortemente la capacità di attrazione degli istituti tecnici e professionali (si veda l'andamento delle iscrizioni), con un allargamento ulteriore del fossato tra capacità dell'istruzione e potenzialità economiche e sociali del Paese. L'articolo 13 stabilisce molto chiaramente che il sistema di istruzione secondaria superiore è un sistema unico, in cui vi è larga parte dedicata all'istruzione tecnica e professionale, e riporta quindi allo Stato questa grande competenza, mentre mantiene naturalmente alle competenze regionali le qualifiche triennali, mettendo in luce i possibili raccordi tra istruzione tecnico-professionale e corsi di formazione professionale, con la valorizzazione dei crediti e la possibilità di raccordi e di relazioni. È molto importante che questo decreto preveda, sempre in questo articolo, il collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa (compreso il volontariato e il privato sociale), con l'università e la ricerca, con gli enti locali. Ricordo che in un importante provvedimento sull'istruzione (la legge che abbiamo che abbiamo approvato in Senato pochi mesi fa sulla riforma degli esami di Stato) vi sono la stessa logica e gli stessi criteri. Questo mettere insieme uno sguardo complessivo sulla legislazione sia del Governo che del Parlamento, sia sull'economia che sull'istruzione, è a mio parere un qualcosa di importante e di notevole per la comprensione della fase che stiamo vivendo. Naturalmente poi vi saranno linee guida appositamente adottate per i raccordi tra questi percorsi. Si tratta ora di mettere i primi pilastri per un disegno che dovrà essere sviluppato e completato nei prossimi mesi. Accanto a questa scelta vi è l'altra, innovativa e altrettanto strategica, dei poli tecnico‑professionali, che comprendono soggetti diversi (gli istituti tecnici e professionali, la formazione professionale accreditata, la formazione tecnica superiore); sono i poli provinciali o subprovinciali, che diventano, nell'area *post*-diploma parallela all'università, la grande area per l'innovazione nelle competenze tecniche e professionali del nostro Paese. Questa è, in un certo senso, una filiera che diventa infrastruttura formidabile per l'Italia, sviluppando le basi della conoscenza e delle competenze professionali utili alla nuova fase dello sviluppo e alle potenzialità e vocazioni dei territori. Naturalmente si richiederà una coerenza interna di sistema in tutto questo e una nuova cultura della scuola secondaria superiore (attraverso provvedimenti che riguarderanno anche i licei, i programmi, gli Una nuova cultura che leghi il grande tema della nuova cittadinanza delle nuove generazioni; penso agli immigrati (e quindi ai temi della interculturalità) che frequentano attivamente le scuole di formazione tecnica e professionale. Tutto questo ha a che fare con una visione complessiva (attendiamo anche il provvedimento per la formazione permanente). In questo quadro, completeremo le indicazioni, la grande scelta politica di questa maggioranza e di questo Governo, per dire che davanti a noi le energie umane e le risorse umane, a tutte le età, sono straordinariamente importanti per la crescita del nostro Paese.

il loro senso di appartenenza e potenzia il ruolo delle istituzioni scolastiche della stessa comunità locale. In questo modo si apre una strada, che va però completata con ulteriori provvedimenti (penso al fondo di perequazione), perché questo

possibilità di prenderne in considerazione il contenuto. Abbiamo la conferma che si sta instaurando un nuovo sistema democratico, per così dire, monocamerale, per giunta

non sia poi così importante vincere. Ebbene, noi siamo diventati tutti decoubertiniani: abbiamo la possibilità di partecipare, ma non solo non vinciamo mai, non lo possiamo perché non ci è dato di competere. Ecco che ci impegniamo in queste belle dissertazioni, piangiamo, ci lamentiamo e critichiamo, ma con l'amara consapevolezza che nulla di quanto diremo potrà cambiare il testo che ci è stato consegnato. Questo non è bello, ma soprattutto

Qui accade come quando a certi bambini si nega quel giocattolo che piace in modo particolare: la reazione isterica è che si rompono anche tutti gli altri giocattoli e non va bene più nulla. In quest'Aula, a volte, si adotta tale atteggiamento. È vero che non tutto è negativo in questo testo, ma dateci la possibilità di dire almeno quello che non va, per poi poter confermare ciò che condividiamo. Come facciamo a non condividere, ad esempio, il provvedimento che riduce i costi fissi e le spese di ricarica nella telefonia mobile? Certamente, vi sono talune disposizioni condivisibili perché vanno - almeno in teoria in teoria - a vantaggio del consumatore. Ma anche qui c'è una lacuna, signor vice ministro Bubbico (visto che è l'unico del Governo che ci ascolta), dacché non vi sono garanzie sul controllo di quest'operazione. Già molti colleghi

Per andare rapidamente sul panorama di tutti gli altri provvedimenti, direi che in generale si realizza una grave ingerenza del Governo nei meccanismi di autoregolamentazione della domanda e dell'offerta sulla base delle più elementari norme di un regime di concorrenza. Non mi strappo i capelli, signor Ministro, per il provvedimento che riguarda la segnalazione dei prezzi dei carburanti in autostrada: esiste già in molti Paesi d'Europa e non è che risolva problemi di carattere democratico, ma soltanto pratico per l'utente. Molto bene, invece, l'intervento sulla trasparenza delle tariffe aeree; noi abbiamo salutato con grande soddisfazione la riforma in questo settore con la liberalizzazione dei servizi aerei che consentirono ad alcune nuove, giovani e avventurose compagnie di contrastare il monopolio delle compagnie nazionali che praticavano - molte lo fanno tuttora - dei prezzi sicuramente fuori dal mercato. Tuttavia, anche in questo caso, l'esortazione fatta a queste compagnie di non indicare prezzi mascherati va controllata e va soprattutto sanzionato

a quell'euro vengono aggiunte le spese aeroportuali e molte altre spese di origini strane: a quel punto non è più una proposta conveniente sul piano del mercato, come le occasioni speciali, speciali, ma diventa una sorta di truffa ai danni del consumatore. Anche in questo caso la legge non indica gli strumenti per controllante ed evitare questa possibilità. Così all'articolo 4, dove si parla di etichettatura di generi alimentari: molto bene la trasparenza nell'obbligo di indicare la scadenza se non fosse per quell'emendamento introdotto alla Camera che consente di smaltire tutte le scorte antecedenti. Quante saranno queste scorte? Come si fa a controllare? Anche qui c'è una lacuna sul piano del controllo. Nel settore dei servizi assicurativi c'è una grave ingerenza e un'altrettanto grave lacuna. Vengono considerate due parti soltanto di questo mercato: la compagnia assicuratrice e l'assicurato, ignorando totalmente la presenza di colui che è l'agente vero del mercato, l'operatore più diretto: l'agente assicurativo, appunto, colui che sta a metà tra la compagnia e il cliente. Non è stato mai ascoltato un rappresentante di questa categoria. Allora è chiaro che molte cose rimangono ancora una volta nebulose, con la compagnia in posizione di forza nei confronti dell'assicurato. Per esempio, sul piano delle polizze poliennali va benissimo l'idea di togliere il vincolo dei dieci anni molte volte l'assicurato meno esperto firma dei contratti senza sapere che in realtà si impegna per dieci anni in maniera irriducibile e che non può più uscire da questo vincolo; giustissimo consentire l'uscita con 60 giorni di anticipo - ma fatelo anche per le polizze inferiori ai tre anni. Mi avvio alla conclusione, Presidente, e quindi all'articolo 13 su cui molti si sono soffermati, il famoso *omnibus* che comprende tutto. Anch'io voglio segnalare la grave ingerenza e non solo nel settore della scuola: qui si butta a mare una riforma molto complessa con quattro emendamenti, come si butta a mare tutto il grande piano delle grandi opere, delle TAV, che nella passata legislatura ottenne l'approvazione dell'Europa. A parte il grave danno economico delle penali che vi saranno da pagare, ritardano sicuramente gli adempimenti che l'Italia deve portare a termine nei confronti dell'Europa. Queste, infatti, non sono opere nazionali, signor Presidente, ma fanno parte di un grande articolato che si chiama TEN (*Trans-European* *Network)*. Se non facciamo noi le interconnessioni, si determinerà una specie di reticolato a singhiozzo, con grave discapito sul piano dei trasporti, dell'economia, ma anche dell'immagine dell'Italia in Europa.

È la liberalizzazione - me lo consentiranno i colleghi - della faccia tosta, una libera possibilità di circolare in quest'Aula con un abbattimento dei costi sul rossore che dovrebbe essere conseguente. Come fa il centro-sinistra, che oggi deve coprire davvero un decreto povero nei contenuti, povero nella metodologia per raggiungere la sua approvazione e povero anche dal punto di vista istituzionale, affrontare con una certa sicumera quelle che dovrebbero essere le pecche dell'opposizione, addirittura richiamando i tempi in cui questa era maggioranza? Come fa il senatore Galardi a dire che le forze del centro-destra non hanno fatto le liberalizzazioni? Intanto mettiamo subito in chiaro un fatto: noi non consideriamo queste delle liberalizzazioni. Sono microinterventi di natura propagandistica che si accaniscono nei confronti - guarda caso - delle fasce più deboli della catena imprenditoriale. Non sono certo i parrucchieri, i panificatori o i distributori della benzina coloro che costituiscono il grosso della costruzione del capitale in Italia e della realizzazione del prodotto interno lordo. Il giorno in cui voi riuscirete a fare una liberalizzazione seria come quella che noi abbiamo dato al mercato del lavoro, il giorno in cui potrete competere con le nostre idee, con la nostra visione liberale del mercato e della società, allora forse il dibattito potrà essere affrontato. Ma oggi con chi parliamo e di cosa parliamo, se siete costretti anche in questa altra nuova microliberalizzazione che definirei la liberalizzazione del dottor cinture elastiche? I vostri stomaci sono diventati particolarmente elastici e direi che la vostra maggioranza si potrebbe ribattezzare non più dell'Ulivo, ma quella del «nonostante». Avrete infatti notato

c'è un «nonostante» che porta i vostri grandi stomaci a digerire porzioni importanti del vostro pensiero, sull'altare del del posto al Governo, sull'altare del non ritorno del centro-destra al potere. Non è così che può continuare. Siamo una delle sette Nazioni più industrializzate del mondo. Questo è il ramo del Parlamento di una delle sette Nazioni più industrializzate e il senatore Cabras vorrebbe affrontare in maniera aperta e libera il tema delle liberalizzazioni. Ma come fate? Non potete, perché siete tanti «nonostante» diversi. Perché, quando parlate delle liberalità a favore delle scuole e di piena attuazione dell'autonomia anche con l'ingresso del capitale privato nelle scuole, non potete farlo ad Aula piena e con il contraddittorio pieno in quanto parte importante, numericamente rilevante della vostra maggioranza su questo non solo non vi segue, ma vi pone anche delle pregiudiziali. Ma «nonostante» si vota il decreto Bersani. E nonostante le tante incongruenze, votate militarmente rinunciando persino a quel minimo di critica che i vostri colleghi alla Camera hanno riconosciuto.

che la disciplina di cui all'articolo 13 fosse stata inserita in un provvedimento normativo specifico. Voi ormai qui al Senato avete persino rinunziato al vostro ruolo di rappresentanti del popolo, di rappresentanti istituzionali sull'altare di quello che deve essere il mantenimento di un Governo che che ormai ogni giorno - è sempre più chiaro - non va verso gli interessi del nostro Paese, un Paese come il nostro che ha grandi sfide davanti. Quindi, parleremo con voi di liberalizzazioni quando vorrete, perché a noi fa piacere parlare, affrontare e decidere su di esse. ciò quando avrete intanto fra di voi le idee chiare e avrete recuperato il senso dell'istituzione e della rappresentanza della volontà popolare. *(Applausi

rispetto a come si è svolto e a come si svolge il dibattito e ai limiti che sono posti al dibattito in quest'Aula. Credo che il problema che viene sollevato sia un problema serio, che riguarda sì la maggioranza, ma anche l'opposizione e credo che insieme dovremo ragionare per fare in modo che le due Aule possano funzionare in modo migliore, con un coinvolgimento maggiore. Ritengo che questa puntualizzazione vada fatta, perché scaricare così le responsabilità dei limiti di un dibattito al Senato solo sulla maggioranza non credo sia giusto. Desidero esprimere il mio apprezzamento per questo provvedimento

hanno introdotto via via nel nostro Paese elementi di liberalizzazione, di tutela e di garanzia per i cittadini. Voglio sottolineare questo aspetto perché ci sono le liberalizzazioni, ma c'è anche una tutela, una garanzia che abbiamo dato ai cittadini. Credo che oggi l'Italia sia un Paese più libero e i nostri cittadini siano più tutelati. È stato fatto un lavoro importante, che sta dando dei frutti e che ne darà in avvenire. Se posso sintetizzare in uno *slogan*, credo che noi ed il nostro Governo abbiamo lavorato per il Paese, per i cittadini e per le imprese,

è una storia antica ed è una storia che molte volte affonda le proprie radici non tanto nella competizione e nella libertà d'impresa, ma nel compromesso con il potere, nella tutela di privilegi, di piccoli e grandi interessi, di patti fatti col potere, sulla scorta dei quali non si sta e non si va in Europa e non si compete con le parti più avanzate dell'Europa. Andare avanti così ci allontanerebbe dall'Europa e ci collocherebbe in serie B; noi invece vorremmo ambire a rimanere in serie A, a giocare nel campionato principale dell'Europa. Anche oggi, così come nel dibattito in Commissione, si dice che si tratta di piccole cose. Io però non credo che si tratti di piccole cose: cose: quando si parla di liberalizzazione o di provvedimenti a tutela e a garanzia del cittadino non ci sono piccole o grandi cose, bisogna affrontarle tutte. In tema di liberalizzazioni e di apertura del mercato, credo che anche le cose più piccole siano importanti. La questione dei farmaci da banco è una piccola cosa?

fino ad oggi ne abbiamo affrontate tante e ne affronteremo altre; ne abbiamo affrontate dal basso, dall'alto, insomma si sta facendo un lavoro complessivo.

Si obietta che le imprese dovrebbero farsi carico di questo; ma io dico un'altra cosa: le famiglie, i cittadini dovrebbero farsi carico di questa tassa impropria, quando l'opposizione si fa paladina del fatto che esiste un Governo che impone solo tasse? In questo caso c'è una tassa impropria e noi proponiamo di abolirla.

su cui tutte le associazioni dei consumatori italiani hanno espresso parere positivo, volto a far risparmiare le famiglie, a conferire nuovo slancio alle imprese, ad accentuare la concorrenza e quindi la vivacità del nostro mercato e a creare trasparenza.

altro che problema di occupazione! Lì non c'era nessun cantiere aperto perché non c'era un euro di finanziamento per la realizzazione di quelle opere.

non si chiude alcun cantiere perché - ripeto - non ce ne sono. Non è partito un solo lavoro da cinque anni a questa parte, cioè da quando

un porto importante nel nostro Paese. Sappiamo tutti quanto la portualità sia una prospettiva di crescita per l'Italia, vista la grande quantità di merci presenti nel Mediterraneo. Si calcola

anzi, ritengo un fatto positivo aver collocato, all'interno di un decreto che ha come obiettivo le liberalizzazioni, la parte riguardante la scuola, ed in particolare quella tecnico‑professionale. Tutti i più attenti analisti e studiosi economici della realtà italiana ci rivelano che, se è vero che ormai la questione del capitale umano è essenziale in tutti i Paesi, perché segna i livelli di produttività e competitività, l'Italia soffre di due problemi: luogo, di scarsa utilizzazione delle capacità da parte del sistema economico-sociale; in secondo luogo di scarsa dotazione di capitale umano. In poche parole, parte, un tessuto economico e sociale che ha difficoltà a valorizzare il merito, perché ingessato in coporativismi e burocratismi, e, dall'altra, uno scarso numero di diplomati e laureati, inferiore a quello di tutti gli altri Paesi europei.

dall'altro, come, attraverso interventi sul sistema dell'istruzione e della formazione, aumentare la nostra dotazione di capitale umano e di capacità.

e la terza «i» era quella di impresa. Bene, il precedente Governo si è concluso con il distacco più grande fra scuola e mondo del lavoro e delle imprese che si sia mai registrato nella storia italiana, con il più vasto fenomeno di licealizzazione cui abbiamo assistito: è diminuita drasticamente la percentuale di iscrizioni nelle scuole di istruzione tecnico-professionale, mentre la stragrande maggioranza delle famiglie ha iscritto i propri ragazzi ai licei.

nei due anni precedenti a questo, le famiglie, quando iscrivevano il proprio ragazzo ad un istituto tecnico-professionale, non sapevano dove lo iscrivevano, nel senso che la sovrapposizione degli ordinamenti, la confusione su chi gestiva e indirizzava questi istituti (lo Stato o le Regioni), la possibilità o l'impossibilità di accesso all'università, questa strana formulazione del liceo tecnologico, che a poco a poco svuotava dei laboratori e della pratica gli istituti tecnici, aveva fatto sì che questo segmento dell'istruzione fosse abbandonato dalle famiglie e, in qualche modo, anche dalle imprese, perché le critiche più grosse al primo impianto del liceo tecnologico della Moratti sono state proprio rivolte da Confindustria e dal sistema delle imprese.

e dell'aumento della capacità dei propri giovani un *asset* fondamentale per lo sviluppo del Paese. La seconda norma introdotta riguarda la questione delle e l'equiparazione del regime fiscale per eventuali donazioni dei privati (famiglie o imprese) alle scuole allo stesso regime delle fondazioni. Sia chiaro che questa è una semplice equiparazione del regime fiscale e che le scuole non diventano fondazioni attraverso questa misura. misura. Credo che questo sia coerente con l'insieme della nostra impostazione; non capisco alcune obiezioni che sono state rivolte anche da settori della sinistra. Ci siamo impegnati perché non si splafonasse nella concessione di soldi pubblici alle scuole private; mi sembra però, a un certo punto, un po' paradossale impegnarsi allo stesso modo perché non vadano soldi privati alle scuole pubbliche,

per evitare che le scuole in situazioni economicamente e socialmente più disagiate avessero dei differenziali di trasferimento molto grandi rispetto alle scuole collocate nei punti di sviluppo. Sulla questione credo che il Governo dovrà porre rapidamente rimedio, perché già oggi le stesse indagini internazionali ci dicono che le differenze di apprendimento, misurate fra i ragazzi italiani, hanno un qualche rapporto con la disponibilità finanziaria delle scuole nelle diverse zone del Paese. Paese. Un istituto tecnico di San Marco in Lamis, per esempio, in Puglia, già oggi, rispetto a un istituto collocato a Prato, a Biella o in Emilia, rileva una differenza di risorse a disposizione per laboratori e attività che è intorno al 30

la scuola potrebbe essere un utile punto di congiunzione tra le imprese e le famiglie, perché è elemento essenziale sia delle politiche per la famiglia sia, se sono vere le cose che ho detto prima,

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come ho già ribadito in questa sede in occasione del mio intervento sul voto di fiducia al Governo Prodi, sono favorevole ad una più profonda e più ampia tutela del consumatore, un impegno del Governo Prodi che ritengo importante e necessario. Allo stesso tempo devo, comunque, nuovamente sottolineare che anche le imprese del nostro Paese, soprattutto quelle medie e piccole, hanno urgentemente bisogno di interventi di sostegno. A tal proposito, accolgo con favore l'articolo 9 del decreto in esame, ossia quello riguardante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Finalmente anche l'Italia fa un passo in avanti, avvicinandosi alle procedure già esistenti in altri Paesi. Tale misura, inoltre, recepisce una direttiva dell'Unione Europea che, nel marzo dello scorso anno, al vertice di Bruxelles, aveva sollecitato gli Stati membri ad interprendere misure tese a far sì che, in tutta l'Europa, un'impresa potesse essere avviata entro una settimana. Tale misura è significativa soprattutto per i giovani che vogliono creare nuove imprese e che, pertanto, hanno bisogno di sostegno e di un clima imprenditoriale favorevole. Favorire l'avvio di una nuova impresa è un primo passo importante, al quale, tuttavia, devono seguire altri provvedimenti tesi a facilitare e semplificare l'*iter* burocratico con il quale le nostre imprese si devono confrontare quotidianamente. Infatti, non è sufficiente semplificare l'avvio di una impresa se, al tempo stesso, un giovane imprenditore deve poi, per puri errori formali, pagare penali altissime. Ribadisco, allo stato ci sono troppi, e spesso del tutto inutili, ostacoli e oneri burocratici che gravano sulle nostre imprese. Pertanto, sollecito fortemente il Governo a ridurre gli stessi. Mi permetto, a tal proposito, di citare nuovamente come esempio la norma che prevede la trasmissione degli elenchi fornitori e clienti, che per gli imprenditori è priva di senso. Bisogna, dunque, intervenire su tali questioni, altrimenti si rischia di scoraggiare fin da subito eventuali nuovi imprenditori. Accolgo positivamente, invece, la modifica introdotta alla Camera dei deputati all'articolo 7 che prevede che l'estinzione anticipata di un mutuo immobiliare non comporti una penale, non solo per l'acquisto della prima casa come previsto nel testo originale -, ma anche per l'acquisto e la ristrutturazione di ogni altra unità abitativa ed immobiliare allo svolgimento della propria attività economica o professionale. Tale misura crea infatti una maggiore competizione sul mercato finanziario e ciò comporta benefici importanti non solo per le famiglie italiane ma anche per i professionisti, per i piccoli imprenditori. Intendo ora porre l'attenzione su una problematica la cui soluzione richiede un maggiore impegno da parte di tutti noi in futuro. Mi riferisco alla tutela del prodotto originale. Quotidianamente veniamo confrontati con prodotti contraffatti, spesso così ben fatti che è difficile persino per un esperto riuscire a distinguere l'originale dalla copia. Si tratta di un problema sentito in tutta Europa, del quale abbiamo discusso a lungo durante l'ultima riunione alla Commissione economica del Consiglio d'Europa. Per fronteggiare questa delicata questione, dobbiamo, insieme agli altri Paesi europei, trovare una soluzione condivisa ed accettata da tutti. Qui, infatti, non si pone soltanto il problema della tutela dell'imprenditore onesto, ma soprattutto quello della tutela dello stesso consumatore. Il consumatore, infatti, deve avere

anche perché non si tratta soltanto di vestiti e di borse ma di prodotti ben più delicati, penso ad esempio ai medicinali. Concludendo, ci troviamo soltanto all'inizio di un processo di modernizzazione. La strada da percorrere è ancora lunga e deve includere, oltre alla tutela del consumatore, anche quella dell'imprenditore onesto.

Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con la conversione del decreto-legge che oggi affrontiamo diamo un segno forte e netto del carattere di questa maggioranza. Troppo spesso si è voluta alimentare l'immagine di una maggioranza rissosa e divisa, oggi ribadiamo invece come sulle questioni concrete, che toccano le condizioni di vita dei cittadini, l'unità e la fermezza di questa coalizione sono salde, e speriamo che questo venga evidenziato. Due elementi innervano questo provvedimento: da un lato, l'idea che la difesa dei consumatori e l'affermazione di nuovi diritti sono scelte non solo giuste ma necessarie alla definizione di un mercato più libero, più equo e più sano; dall'altro, l'idea che l'eliminazione di vincoli di sapore feudale possa offrire nuove opportunità di autonomia per i cittadini e per i giovani in particolare. Quella di oggi è la tappa di un percorso avviato poco dopo l'inizio della legislatura e che sono convinto ci accompagnerà fino alla conclusione di questo percorso, che io spero di cinque anni. Taxi, energia, gas, farmaci, supermercati, assicurazioni, mutui, ipoteche, conti correnti, prodotti alimentari, estetiste e guide turistiche, ricariche telefoniche, autoscuole, autoscuole, sono alcuni dei tanti comparti che in soli dieci mesi sono stati toccati da interventi di liberalizzazione. Si tratta di interventi che cambiano concretamente la vita delle persone, che ne definiscono il futuro. ad un giovane, ad esempio, che dopo aver passato anni a tagliare i capelli nel proprio appartamento, al nero, oggi ha la possibilità di aprire un proprio negozio, di costruire un percorso autonomo, di cercare di cambiare la propria vita. Stiamo offrendo piccole ma concrete opportunità a tutti e tutte. Si pensi ai lavori pieni di fatica e dignità, come i compiti di facchinaggio e pulizia. Con questo decreto ci saranno più possibilità e più occasioni anche per i più deboli. Alcuni commentatori in questi mesi si sono appassionati a dire che si trattava di poca cosa e che i problemi sono ben altri. Francamente, ritenere che la restituzione di alcuni miliardi di euro alle famiglie - che ha il sapore di risarcimento - attraverso la riduzione di spese improprie o cavillose o la riduzione del costo della vita, per tanti cittadini sia poca cosa è segno di una fastidiosa superficialità. Le ricariche telefoniche, che tanti motti di spirito hanno prodotto, significano solo nel 2005 più di un miliardo di euro, come è stato ricordato, sottratti alle disponibilità delle famiglie. Così come gli interventi sui mutui e sulle assicurazioni hanno degli effetti immediati e concreti nel garantire diritti fondamentali come il diritto alla casa. Assicurare la portabilità dei mutui e riportare ad equità le penali per estinzione anticipata sono provvedimenti importanti, soprattutto in un momento in cui il basso costo del denaro, da un lato, e la corsa all'acquisto dall'altro, hanno reso estremamente oneroso comprare una casa. Anche qui non si tratta di poca cosa. Di fronte a prezzi immobiliari come quelli cui assistiamo nelle aree metropolitane, e non solo, qualunque intervento capace di ridurre il carico delle famiglie si rivela quanto mai urgente. Citiamo solo qualche numero. Secondo i dati della Banca d'Italia un terzo del reddito di una famiglia serve a pagare il mutuo per la casa e per le fasce deboli si arriva al 40 per cento. Per acquistare invece una casa nel 1965 bastavano tre annualità di stipendio, nel 2004 ne servivano nove, il triplo. Di fronte a questo scenario è evidente come una maggiore concorrenza agevolata dalla portabilità dei mutui, e quindi un abbassamento dei tassi di interesse, sia uno fattore di grande impatto sociale. Questi temi, quindi, dai mutui alle ricariche, non solo rendono il nostro sistema più competitivo e libero, ma consentono anche di abbattere il costo della vita e di restituire risorse importanti ai cittadini. In queste settimane, di fronte al miglioramento delle entrate si sta molto discutendo della destinazione degli 8 miliardi aggiuntivi che l'impegno contro l'evasione fiscale e la crescita del Paese hanno prodotto e alcuni hanno sollecitato una riduzione del carico fiscale, che è sicuramente un obiettivo su cui riflettere con attenzione. Ma è necessario avere anche la consapevolezza che la leva fiscale non è l'unica che ci consente di ampliare la disponibilità delle famiglie: un mercato chiuso, dove troppi costi sono irragionevoli, dove posizioni monopolistiche o di cartello possono lucrare sui prezzi; sono anche essi pesi che gravano ingiustamente sui redditi. Proprio perché questi interventi raggiungono il duplice fine di costruire un sistema di mercato più competitivo e di alleggerire le spese a carico delle famiglie, non capiamo i motivi dell'atteggiamento cui abbiamo assistito alla Camera da parte dell'opposizione, un atteggiamento che ora pesa grandemente sui nostri lavori, visto che in una settimana dobbiamo convertire il decreto, quando l'altro ramo del Parlamento ha impiegato quasi 50 giorni per trasmetterlo al Senato. Non capiamo quel l'atteggiamento perché avremmo sperato di essere sfidati sul terreno di più ampie e più forti liberalizzazioni e abbiamo assistito invece a un gioco al ribasso e alla difesa di interessi corporativi contrari all'interesse generale. La dialettica parlamentare tra maggioranza e minoranza può essere una grande occasione per rafforzare le scelte proprio nell'interesse generale e credo sia chiaro che riteniamo sbagliata l'idea di un bipolarismo tra sordi. Purtroppo dobbiamo registrare come la dinamica che ha portato questo provvedimento al Senato non sia stata questa e che oggi non abbiamo tempo di introdurre miglioramenti al testo. Nel corso della legislatura avremo sicuramente altre occasioni, signor Ministro, per costruire un percorso largo, che consenta di fare del nostro Paese un Paese più europeo, dove tra il binario che tiene insieme merito e concorrenza e quello che invece vede, da una parte, il clientelismo e, dall'altra, la burocrazia possa compiere sicuramente una scelta chiara e profonda da parte nostra. Noi sceglieremo sempre quel binario che tiene insieme il merito e la concorrenza. A partire dal disegno di legge già licenziato dal Consiglio dei ministri sempre in materia di liberalizzazioni abbiamo ancora molta strada da fare. Mentre noi intraprendiamo questo percorso anche l'Europa si muove; dovremo essere rapidi a portare il nostro Paese al livello dei *partners* europei. Pensiamo ad esempio all'impatto benefico che la direttiva sui sistemi di pagamento, ora in discussione a Bruxelles, potrà avere sul nostro mercato. Sono tutti interventi profondi e efficaci e quindi sarà necessario gestire la fase di transizione con la giusta flessibilità e assicurare un rigoroso controllo sugli effetti delle norme che andiamo ad introdurre. Per questo sarà determinante la riuscita della trasmissione telematica, che consente di accelerare i tempi di controllo. Presto affronteremo, sicuramente con tempi più distesi, il pacchetto contenuto nel disegno di legge ora all'esame della Camera e, oltre a queste misure, che convertiremo in legge nella seduta odierna, restano aperte alcune scelte che non sono state ancora affrontate. Ne cito a titolo di esempio solo alcune. La prima è il mercato dell'informatica e del *software*, dove vigono, soprattutto nei sistemi operativi e nei prodotti da ufficio posizioni dominanti che frenano il mercato. L'incompatibilità di formati e di modelli commerciali che obbligano di fatto all'acquisto di *hardware* e *software* congiuntamente tendono a confermare questa posizione. Una competizione fondata sulla qualità del prodotto e sul prezzo consentirebbe di abbattere il prezzo dell'acquisto di un PC, invece di rincorrere nel corso degli anni le detrazioni fiscali. La seconda è la necessità di una liberalizzazione vera sulle piccole fonti di energia rinnovabili destinate all'autoconsumo. Grazie al decreto che votiamo oggi sarà possibile aprire un'impresa in un giorno; ma un normale cittadino, per avere l'allaccio del proprio impianto fotovoltaico o a biomasse, deve ancora aspettare alcuni mesi. E questo, anche di fronte agli sforzi che il Governo sta compiendo per promuovere le fonti rinnovabili, non è accettabile; bisogna intervenire e semplificare. Un terzo esempio - ed è l'ultimo - sono gli strumenti di tutela dei consumatori, come la *class action*. Se si assicurano nuovi diritti ai consumatori, devono essere garantiti anche adeguati strumenti per rendere questi diritti cogenti; il ricorso collettivo è il primo e più forte strumento per spingere le imprese a rispettare pienamente queste nuove tutele. anche dopo i risultati che con la conversione del decreto riusciremo a raggiungere, resta di fronte a noi una grande sfida e una lunga strada. Cresce la domanda da parte dei cittadini, crescono le aspettative. E noi non abbiamo nessuna intenzione di deluderli.

la misura della decretazione d'urgenza su questi argomenti, anziché affrontarli con il dovuto tempo per ogni singolo argomento, sia stato utile

la trasparenza e la libertà di recesso dei contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi Internet. Ciò, in sostanza, ci vede abbastanza d'accordo. Mi pare che l'abolizione dei costi di ricarica sia sicuramente un intervento dovuto, anche se qualcuno dice che che non era il caso che se ne occupasse il Governo. Io dico invece che va bene che qualcuno se ne occupi; bisognava affrontare però, al contempo, quella che è la realtà. Già alcuni organi di stampa stanno affrontando l'argomento e dicono che non ci sarà nessun utile a favore dei cittadini. Non so se questo sia vero, non ho fatto i conti. letto invece - e vado a leggere - l'intervento del sottosegretario Lettieri in V Commissione alla Camera. Ad una precisa richiesta di chiarimento (se l'articolo 1 comportasse o meno un minor gettito finanziario, in quanto l'abolizione dei costi di ricarica avrebbe determinato una diminuzione del fatturato),

o del panettiere, ma se c'è un minore esborso per i cittadini, ci deve essere - di conseguenza - anche una minore entrata per le compagnie.

che durano da quasi 20 anni e nessuno ha mai detto niente o è intervenuto. Non è tutela dei consumatori far sì che queste liquidazioni abbiano una minor durata? Credo che si sia persa una grossa occasione, oppure l'ISVAP è uno dei quei carrozzoni intoccabili?

di quella tutela dei consumatori che voi sbandierate nella presentazione del vostro provvedimento.

imprese che nei Paesi europei e nei Paesi al livello di economia mondiale si riesce ad aprire in due o tre giorni.

Sull'articolo 10, riguardante la liberalizzazione delle piccole attività, e cioè parrucchieri, barbieri, estetisti, eccetera, abbiamo pressioni da parte delle autoscuole che non so se ritenere giuste o sbagliate. Molto probabilmente,

Sappiamo che le cooperative, tra la grande distribuzione, sono quelle che hanno una fetta maggiore del fatturato, perciò se qualcuno attraverso questi interventi vede un certo favore verso la grande distribuzione non ha tutti i torti, anche perché quella norma che prevede che la grande distribuzione possa vendere prodotti assegnati alla "Esso" - cito, per esempio, le benzine ma potrebbero essere anche i prodotti farmaceutici - dovrebbe vedere la reciprocità della cosa.

di essere il più sintetico possibile affrontando l'argomento più importante, quello che è stato più dibattuto: mi riferisco alla revoca delle concessioni TAV. Io credo che un articolo del genere, in uno Stato di diritto - e spero di essere smentito su questo - non sia fattibile. Si è parlato di incostituzionalità; non voglio assolutamente confrontarmi con costituzionalisti ed esperti del settore, ma anche il buonsenso mi dice che non si può andare contro ad un diritto acquisito. Non so se si risparmia o meno. So di sicuro che ci sono degli sperperi di risorse, risorse già impiegate, che qualcuno ha quantificato in 20 miliardi di euro. Non

Questa era una cosa troppo grave, troppo importante, troppo fuori dalle righe - se mi si passa la parola - per essere affrontata in un decreto-legge di questa vastità.

un atteggiamento di completa chiusura e di completa contestazione. In conclusione, signor Ministro, ringraziandola per l'attenzione, che avremmo veramente voluto che ci fosse quella collaborazione fra maggioranza e opposizioni per argomenti di tal genere che di politico - a mio a mio avviso - hanno poco ma sono veramente - lo riconosco - sopra le parti politiche. La tutela dei cittadini, la tutela della trasparenza, la tutela del consumatore non può essere assolutamente una questione politica ma può essere veramente una questione *bipartisan*. Abbiamo perso una grande occasione perché ciò avvenga.